con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Vorrei esprimere, a nome mio personale e dell'Assemblea, un bentornato al senatore Calderoli.

senatori, lo scorso 24 gennaio ricorreva il 40° anniversario dell'assassinio di Guido Rossa, operaio, sindacalista e militante del Partito Comunista Italiano. Ho sinceramente apprezzato l'invito, formulato da alcuni senatori nel corso dell'ultima seduta, di dedicare l'inizio dei lavori odierni al ricordo di un uomo di grande generosità e coraggio, un lavoratore che aveva a cuore le condizioni dei colleghi, per i quali si era sempre battuto con tenacia e determinazione. Aveva iniziato a lavorare in fabbrica giovanissimo, a quattordici anni. Aveva una famiglia che amava e alla quale è stato brutalmente strappato dai colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui in quella fredda mattina del 24 gennaio 1979. Fu una vera e propria esecuzione. In uno dei momenti più drammatici della storia del nostro Paese, mentre la paura inibiva le coscienze e il terrore paralizzava le persone, Guido Rossa, con la naturalezza di chi crede fermamente nella legalità, aveva denunciato un collega che, nella fabbrica dove lui lavorava, fiancheggiava e collaborava con i brigatisti. Fece il suo dovere da cittadino, da uomo giusto, da uomo libero. Guido Rossa, in questi quaranta anni, ha rappresentato il simbolo della fermezza contro l'odio del terrorismo. Era una persona per bene, non voleva essere un eroe. Eppure fu un eroico esempio di senso civico e di rispetto per la giustizia; un cittadino esemplare che quest'Aula e il Paese tutto hanno il dovere di commemorare affinché anche le future generazioni sappiano che, persino nei momenti più difficili della Repubblica, c'è stato chi ha consapevolmente scelto di difendere i valori del nostro Stato di diritto. Come ha saggiamente ricordato il Presidente della Repubblica, non si può costruire un futuro di pace e di armonia se non si preserva la memoria delle violenze e degli anni più bui del nostro passato.

il decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 giunge in Aula dopo una lunga istruttoria nelle Commissioni riunite affari costituzionali e lavori pubblici. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame nelle Commissioni hanno ampliato il contenuto del provvedimento, apportando notevoli migliorie al testo e soprattutto semplificazioni per i cittadini e le imprese. Permettetemi di ringraziare innanzi tutto gli uffici delle Commissioni riunite 1a e 8a per il sempre prezioso supporto e l'esemplare pazienza dimostrata nel corso delle lunghe giornate

Venendo ai contenuti, il decreto-legge semplificazioni reca disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione volte a superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche del rapporto di mercato e con la pubblica amministrazione, nonché criticità riscontrate nella realtà sociale quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 1 (emendamento 1.44 (testo 2)) istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale, con dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, a valere sulle disponibilità vigenti del Fondo, dedicata a interventi di garanzia a condizioni di mercato in favore di piccole e medie imprese che siano in difficoltà nella restituzione delle rate di un finanziamento precedentemente contratto con banche o intermediari finanziari, classificato come «inadempienza probabile» nella centrale rischi della Banca d'Italia, e che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sezione speciale del Fondo interviene per rilasciare una garanzia alla banca o all'intermediario che ha erogato il prestito per il quale l'impresa ha incontrato difficoltà di restituzione. La garanzia cessa con l'avvenuto pagamento del credito certificato da parte della pubblica amministrazione ed è subordinata alla sottoscrizione - tra la banca o l'intermediario finanziario e la piccola e media impresa beneficiaria - di un piano di rientro di durata massima di vent'anni. La garanzia copre - nella misura indicata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro - il minore tra l'importo del finanziamento non rimborsato dalla piccola e media impresa maggiorato di interessi e l'ammontare del credito certificato. Gli interventi di garanzia sono estesi anche ai professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi. L'efficacia del regime di aiuto è condizionata alla preventiva notificazione della Commissione europea. L'articolo 3 sopprime la previsione che disponeva la tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro presso il Ministero del lavoro a partire dal primo gennaio 2019 e che demandava a un decreto del Ministro del lavoro - mai emanato l'individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro. 8-*ter*, ridefinisce i termini dell'entrata in vigore del comma 51 della legge n. 145 del 2018, che prevede l'abrogazione delle agevolazioni tributarie definite per specifiche categorie di soggetti (tra i quali, enti di assistenza sociale, istituti di istruzione e istituti autonomi per le case popolari). L'entrata in vigore viene subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi che individuino nuove misure di favore nei confronti di soggetti che realizzano finalità sociali. Il comma 34 dispone che la tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni materiali strumentali e per l'assunzione di personale, di cui ai commi da 28 a 33, sia cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito. L'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del prestito erogato ad Alitalia sulla base del decreto-legge n. 50 del 2017, che sarebbe dovuto scadere il 15 dicembre 2018. Il nuovo termine è fissato al trentesimo giorno dalla data in cui acquisterà efficacia la cessione dei complessi aziendali facenti capo alla società in amministrazione straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2019. L'articolo 3, comma 1-*bis*, interviene sulla platea dei destinatari del Programma nazionale triennale della pesca. In particolare, esso inserisce tra i destinatari del Programma nazionale triennale della pesca, relativamente alle iniziative di promozione della cooperazione e dell'associazionismo e a favore dei lavoratori dipendenti, anche le associazioni nazionali delle imprese di pesca stipulanti il CCNL di riferimento del settore. L'articolo 3-*bis* (emendamento 3.0.8) apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo. In particolare, si vieta di far agire nei locali di proprietà nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità. L'articolo 3-*bis* (emendamento 3.0.81 (testo 3)) amplia il lasso temporale (portandolo da tre a ventiquattro mesi) entro il quale il datore di lavoro che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non sia punibile né assoggettabile a sanzione amministrativa. L'articolo 3-*bis* (emendamento 3.0.136 (testo 2)) inserisce una serie di agevolazioni per le imprese che operano nella zona logistica semplificata

L'articolo 3-*bis* (emendamento 3.0.500) affida all'AGEA il compito di avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, a un unico fornitore, della gestione ed evoluzione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fermi restando gli effetti e l'ulteriore corso dei lotti già assegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. L'articolo 3-*bis* (emendamento 3.0.700) rende obbligatorio riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l'indicazione del luogo di origine in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti. L'articolo 4, comma 2 (emendamento 4.3 (testo 3)) interviene sull'articolo 560 del codice di procedura civile, garantendo al debitore e ai suoi familiari conviventi il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare. L'articolo 4-*bis* (emendamento 4.0.1000) prevede la corresponsione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime del disastro avvenuto presso l'hotel «Rigopiano» di Farindola, in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, e per coloro che siano stati gravemente feriti. L'articolo 5 interviene sul codice dei contratti pubblici, apportando una modifica all'articolo 80 - relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o di concessione al fine di renderne la formulazione maggiormente conforme alla corrispondente disposizione della direttiva europea sugli appalti. L'articolo 7 amplia in via transitoria - dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020 le competenze del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (DAP), al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso. L'articolo 9*-bis* (emendamento 9.0.41 (testo 2)) demanda a un decreto ministeriale la definizione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale affida a un Comitato paritetico la proposta di ridefinizione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale; definisce i casi in cui la Regione è considerata adempiente agli obblighi di contenimento delle spese di personale e impone alle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari o ai piani operativi obblighi in materia di revisione degli obiettivi di spesa del personale. L'articolo 9*-bis*, comma 1 (emendamento 9.0.500 (testo 2)), detta alcune disposizioni in tema di personale del Servizio sanitario nazionale, modificando alcune norme della legge di bilancio per il 2019. I commi da 360 a 366 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 concernono le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime. Il comma 687 prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, rimanga nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione, nei termini previsti dalla medesima, della delega relativa alla riorganizzazione e, in particolare, al nuovo inquadramento della dirigenza pubblica. L'articolo 10*-bis* (emendamento 10.0.1000) introduce disposizioni in materia di servizio di noleggio con conducente e alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio, prevedendo che la richiesta del servizio NCC possa essere effettuata presso la sede, oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici; si richiede che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o Area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. È prevista una disciplina derogatoria per le sole Regioni Sicilia e Sardegna. Con riguardo a tali Regioni, l'autorizzazione rilasciata in un Comune della Regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa. (testo 3)) reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo l'approvazione di un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI), volto a offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, nella valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. (testo 3)) interviene sulla disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il nuovo comma 1 stabilisce che, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico passano, senza compenso, in proprietà delle Regioni, in stato di regolare funzionamento. L'articolo 11-*bis* (emendamento 11.0.1000) reca una disposizione di interpretazione autentica volta a ovviare alle incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. La disposizione, inoltre, contempla una proroga di sei mesi per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018. (testo 2)) reca misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali relative alla posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni; al differimento al 28 febbraio del termine riguardante determinati adempimenti a carico degli enti locali; all'ampliamento della possibilità di contrarre mutui, anche per gli enti in dissesto, per finanziare le spese di investimento strettamente funzionali ai progetti e interventi cofinanziati dall'Unione europea o da altre amministrazioni o enti, pubblici o privati;

all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali; all'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari; alla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; al riparto in cinque annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro; alla proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali; all'incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo attribuito ai Comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI, nonché alla quantificazione e copertura dei relativi oneri finanziari; al contrasto di fenomeni fraudolenti in materia di IVA nell'ambito di transazioni commerciali di determinati beni elettronici effettuate tramite piattaforme commerciali *online*; al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo di 190 milioni di euro, *ex* articolo l, comma 845, della legge di bilancio 2019;

all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009 relativa all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano, che gli esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità chiamati a integrare la composizione dell'Osservatorio devono essere comunque pari a cinque.

il presidente Coltorti ha già fatto un esame molto dettagliato dei contenuti del

e devo dire che abbiamo trattato talmente tanti aspetti che siamo stati anche redarguiti per il fatto che forse abbiamo lavorato troppo. Sentirmi dire che abbiamo lavorato troppo e che abbiamo fatto troppe cose non può che far piacere non solo a me personalmente, ma parlo per tutta la maggioranza di Governo. Penso anche

troppo importanti: mi riferisco ad esempio alla questione del codice degli appalti. Quello che è giusto che sappiano i cittadini e le associazioni di categoria è che i temi che non sono stati trattati e che non saranno esaminati oggi

infatti scontato quanto è stato detto rispetto al rapporto che si è tenuto nel corso dei lavori delle Commissioni. Per quanto ci riguarda, come Gruppo Partito Democratico abbiamo seguito la nostra cultura politica, quindi abbiamo messo in campo la nostra esperienza, la nostra intelligenza, ma soprattutto il rispetto per i diversi ruoli che ognuno di noi esercita all'interno del Senato della Repubblica: chi ha il dovere di governare e chi ha il diritto-dovere di controllare e di fare le proprie proposte. Per quanto riguarda, invece, il merito del provvedimento, se il decreto-legge in esame intendeva superare situazioni di criticità che rilevo dal titolo (le dinamiche dei rapporti del mercato con la pubblica amministrazione, le criticità riscontrate nella realtà sociale quale il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza dei medici di medicina generale, e così via), siamo convinti che questi obiettivi, pur lodevoli, non siano stati raggiunti, anzi possiamo dire che vi è un fallimento rispetto all'obiettivo iniziale. Questo perché non solo non si colgono le soluzioni, ma perché il decreto-legge è stato di fatto stravolto con una serie di emendamenti, che solo in parte sono stati respinti per inammissibilità o ritiri spontanei dopo cruente contrapposizioni all'interno della maggioranza che hanno ritardato non poco la conclusione dei lavori delle Commissioni Nell'assalto che c'è stato, fanno certamente rumore alcuni aspetti, rispetto alla propaganda che abbiamo sentito in questi mesi. sono cioè delle proposte che sono esattamente il contrario di quanto è stato ripetuto in ogni dove nel nostro Paese. Ne elenco alcune, in modo che gli italiani possano comprendere bene la differenza con la realtà. Ad esempio, è stata curiosa la decisione di acquistare quote della Banca europea degli investimenti; si tratta di una banca particolare, ma è pur sempre una banca, peraltro dell'odiatissima Europa: questa inversione di tendenza ovviamente a noi non può che far

Colpisce poi quel mirato emendamento *ad personam*, che incarica il commissario straordinario per Genova, il sindaco della città, a scegliere quello che riteniamo un certo e ben conosciuto operatore della logistica (lo ritroveremo poi nell'emendamento). l'esilarante inno ad Equitalia, sempre avversata, ma che avete deciso di potenziare, per incrementare le entrate all'erario del Paese. Vanno poi rilevati il favore che fate agli odiatissimi concessionari autostradali, nel momento in cui concedete una deroga fino a dicembre di quest'anno per l'applicazione del codice degli appalti, oppure la pericolosa deroga all'adeguamento degli impianti antincendio nelle scuole italiane: si prevedono ancora tre anni per adeguarsi. finanziare il reddito di cittadinanza, togliete soldi alla sicurezza dei nostri figli. Va poi ricordato il favore che fate alle assicurazioni, contro gli interessi degli assicurati, che saranno costretti a subire ulteriori costi nel momento in cui dovranno disinstallare le scatole nere ad ogni cambio di assicurazione.

un risultato evidente della nostra azione politica e della nostra contrarietà. In sincerità, è stato assurdo anche solo pensare tale norma e, quindi, il fatto che vi sia stato un ripensamento da parte della maggioranza, che certamente ridarà serenità all'intero comparto, è un fatto che abbiamo apprezzato e che è in linea con quel rapporto corretto che abbiamo stabilito nei lavori della Commissione. Dunque, al termine del lavoro della Commissione è emerso un prodotto deforme rispetto alla volontà iniziale, anzi, come anche altri colleghi hanno evidenziato - in particolare il collega Schifani - si pone una seria valutazione sullo stravolgimento successivo di un decreto-legge rispetto alla volontà iniziale. un fatto che, in casi simili, in passato, è stato già stigmatizzato dalla Corte costituzionale. Auspichiamo che ci sia anche in questa tornata una valutazione della Presidenza, perché va bene il richiamo alle regole per tutti, ma poi, nel momento in cui vengono avanzate proposte che nulla hanno a che vedere con il testo originario, come molti degli emendamenti presentati, si pone un problema di rispetto delle prerogative, non solo della Presidenza, ma anche di quanto stabilito dalla Corte costituzionale. nel merito, l'articolo 1, come noto, istituisce, nell'ambito di un Fondo di garanzia già esistente per le piccole e medie imprese, una sezione speciale, con una dotazione di 50 milioni di euro, a valere su tale disponibilità,

fronteggiare le difficoltà che realmente esistono nel Paese, ma non riteniamo comprensibili alcune delle scelte conseguenti per rispettare questa idea. Evidenzio queste esigenze, ponendo alcune domande, che poi sono state oggetto dei nostri emendamenti: perché per colui che è in difficoltà nella restituzione delle rate di un finanziamento, che ha contratto con un istituto bancario o con una società finanziaria, e che è anche titolare di crediti certificati nei confronti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, si è deciso l'intervento della sezione speciale per rilasciare una garanzia alla banca? Perché questo difficoltoso meccanismo a favore, ovviamente, di coloro che sono in difficoltà? Perché ulteriori orpelli burocratici, il piano di rientro ventennale e i costi relativi, e non invece consentire alle persone e alle piccole e medie imprese in difficoltà di pagare le rate del finanziamento, che ha determinato, peraltro, la sofferenza probabile, con lo stesso credito maturato con la pubblica amministrazione? Non sarebbe stato più lineare? In questo In questo modo si sarebbe anche superata quella che noi riteniamo l'assurda contraddittorietà del sollievo economico che il Governo vuole garantire, ovvero solo fino all'80 per cento del minore tra l'importo del finanziamento non rimborsato dalla piccola e media impresa e l'ammontare del credito certificato. Abbiamo presentato una proposta su questo particolare passaggio ma, com'è noto, non l'avete accolta e l'avete bocciata. La possibilità di accedere alla nuova sezione specializzata del fondo di garanzia è stata limitata alle piccole e medie imprese. È un restringimento che riteniamo ingiustificato perché esclude dal beneficio previsto le microimprese che oggi possono liberamente accedere al fondo di garanzia. Fortunatamente, grazie ad uno degli emendamenti che abbiamo presentato, la maggioranza ha inserito tra i beneficiari anche i professionisti, quindi un correttivo è stato apportato, sebbene non esaustivo rispetto alla platea delle persone e delle imprese in difficoltà. E perché le imprese del settore edile non possono avere accesso alla sezione specializzata del fondo di garanzia? Per quale ragione, a parità di oggetto, che è poi il credito verso la pubblica amministrazione, sono stati decisi trattamenti diversi? Noi avevamo proposto di inserirle tra i beneficiari, ma la cosa non è andata in porto. Altrettanto avete fatto con la qualificazione del fondo: com'è noto, l'assegnazione nella sezione speciale di 50 milioni di euro non copre praticamente nulla. I crediti per le imprese e i debiti per la pubblica amministrazione sono ben altri, quindi il rischio è che non tutti coloro che sono in difficoltà e che hanno crediti nei confronti della pubblica amministrazione potranno aderire alle previsioni favorevoli della sezione speciale del fondo di garanzia. Per questa ragione, avevamo presentato un emendamento per incrementare quel fondo, ma questo emendamento è stato bocciato. Abbiamo posto il tema del dissesto degli enti locali: locali: noi ritenevamo e riteniamo ancora oggi che coloro che hanno crediti nei confronti degli enti locali in dissesto, che sono difficilmente esigibili, debbano avere una priorità nell'accesso alla sezione speciale del fondo di garanzia, ma la nostra proposta non è stata accolta ed è stata bocciata, come pure

quale quello delle imprese che sono in conclamata difficoltà ma non hanno crediti nei confronti della pubblica amministrazione e sono completamente escluse da qualsiasi tipo di beneficio, come pure quello di tutte le imprese che hanno subappalti nei confronti di imprese, che invece sono in difficoltà economiche e hanno crediti verso la pubblica amministrazione. Queste imprese sono le prime a saltare e infatti purtroppo, nonostante un nostro emendamento in questa direzione, non sono state comprese tra i beneficiari della sezione speciale del fondo di garanzia.

per rasserenare e consentire la continuità aziendale. Adesso, però, tocca dare seguito a tutte le azioni che allora avevamo immaginato, nel momento in cui è stato concesso quel prestito, per dire che le scelte che bisogna fare su Alitalia bisogna farle in fretta e a breve termine, altrimenti avremo il rischio, tra non molto, di derogare ancora la restituzione del credito. Quindi basta con le proroghe: occorre accelerare la definizione di un percorso che dia un futuro certo alla nostra compagnia di bandiera, ma su questo ci misureremo nei prossimi mesi. Con l'articolo 3, che supera - sopprimendola, purtroppo - la modalità telematica del Libro unico del lavoro presso il Ministero del lavoro è stata compiuta, a nostro modo di vedere, un'oscenità. Ritenere infatti che questa tenuta digitale non sia utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, così com'è scritto nella relazione che accompagna il provvedimento, è rinunciare ai compiti che i due enti, Ministero e Ispettorato, devono svolgere. Devo ricordare all'Assemblea che il Libro unico del lavoro aveva sostituito il libro matricola e il libro paga, che ogni datore di lavoro privato doveva tenere: rinunziarvi significa tornare indietro di molti anni e consentire di brindare a coloro che invece di quei libri hanno fatto di tutto,

Voglio qui ricordare la richiesta di estendere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali spettanti ai coltivatori diretti anche ai mezzadri coloni, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari soggetti soggetti all'obbligo di assicurazione per invalidità e vecchiaia. Voglio qui ricordare inoltre la proposta di prorogare l'entrata in vigore della revisione delle macchine agricole, in attesa di conoscere la tipologia delle verifiche da effettuare in sede di revisione,

della famosa ecotassa sulle auto, fintanto che un tavolo tecnico-politico, con la partecipazione di diversi soggetti, che poi vedremo, non definisca linee guida per l'acquisto di veicoli elettrici di nuova fabbricazione.

le lesioni gravi stradali a querela di parte, anziché come accade adesso. Si tratta di un'assurdità, che ha fatto pensare ad un intervento mirato nei confronti di qualche situazione di difficoltà nel nostro Paese. Pensiamo che deflettere sulla gravità di tutto quanto concerne gli incidenti stradali sia inaccettabile e, per fortuna, quest'aspetto è stato ritirato anche grazie alla nostra ferma contrarietà.

Rispetto all'iniziale intenzione di modificare il codice degli appalti, deregolando il settore, vi è stata un'intelligente decisione, da parte della maggioranza, nel dibattito che ha avuto luogo all'interno all'interno della Commissione. Abbiamo apprezzato la volontà di fare in modo che tutta la discussione riferita al codice degli appalti sia dedicata in un procedimento specifico, quale potrebbe essere quello annunciato, ossia la legge delega. in questa direzione, non faremo mancare il nostro contributo. A questo proposito, però, potevate risparmiarvi alcune considerazioni contro l'autorità anticorruzione e, in particolare, contro il presidente Cantone.

attribuendoci posizioni sempre migliori nella classifica dei Paesi meno corrotti al mondo, qui ci interroghiamo se la difficoltà del blocco degli appalti pubblici sia causata dall'impegno del presidente Cantone e dell'ANAC e, addirittura, dal codice degli appalti. Temiamo che i motivi siano altri, se questa è la vostra intenzione. che, dietro le pur legittime considerazioni e possibili correzioni del codice degli appalti, si nascondessero appetiti diversi, come un ritorno al passato, come purtroppo confermano alcune delle vostre proposte approvate nella legge di bilancio. Ci sono poi degli aspetti che noi riteniamo fondamentali, su cui abbiamo proposto di intervenire, ma la nostra proposta l'abrogazione della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, un mostro a cui ancora oggi, dopo un mese, non sono stati attribuiti il *nomen*, l'allocazione, l'organizzazione e le funzioni. Lo ritiriamo un inutile orpello burocratico neocentralista, che, secondo voi, dovrebbe favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione. Noi non crediamo che serva un elefante simile. Sarebbe bastato lasciare Casa Italia, la struttura di missione che avete ideologicamente cancellato e che raggiungeva gli stessi obiettivi che vi ponete, ma con un metodo diverso, che è quello che serve. Il problema non è quello di effettuare la progettazione, ma di superare tutte le difficoltà. Servono pertanto un coordinamento tra enti, una *moral suasion*, una funzione politica e la risoluzione dei conflitti. Non serve una progettazione in quella direzione. Abbiamo poi chiesto di cancellare la decisione di elevare il limite, per effettuare una gara pubblica, da 40.000 a 150.000 euro, perché pensiamo che una decisione del genere debba rientrare nell'ambito della più articolata riflessione che si vuol fare per quanto riguarda il codice degli appalti. Farlo in un contesto scollegato come quello della legge di bilancio o come questo, come sta avvenendo, e senza controbilanciamenti può rischiare di favorire appetiti che il codice degli appalti voleva invece

È stato eliminato un sistema di tracciabilità dei rifiuti che, seppur con mille problemi perché faceva emergere tante problematiche, non può essere sostituito, nemmeno temporaneamente, con ciò che lo stesso SISTRI aveva superato. di un vero colpo di spugna, che pensiamo ci riporti indietro negli anni, a un'epoca che ha segnato e devastato interi territori del nostro Paese, in del nostro Paese, in particolare nel Mezzogiorno, dove sono state sversate in modo incontrollato tonnellate di rifiuti nocivi di origine industriale. Conosciamo bene le difficoltà del mondo delle imprese rispetto alla complessità di questo meccanismo. Tuttavia, le difficoltà non si superano cancellando il meccanismo e tornando indietro, perché così si fa peggio.

maniera indisturbata. Ci è stato detto che adesso l'obiettivo è quello di inserire un nuovo sistema di tracciabilità e noi speriamo che il Governo agisca in fretta, con nuove modalità. Ma se i tempi saranno lunghi, che senso ha avuto cancellare il SISTRI? Non sarebbe stato meglio tenerlo in piedi, anche se con difficoltà? Altrimenti, si chiarisce bene quali siano stati gli obiettivi della cancellazione di questo importantissimo strumento.

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la costituzione di una società. Consideriamo questo un errore concettuale, come se il problema di questo settore fosse la gestione e non il fatto che servono risorse. Anziché fare questo tipo di struttura - l'ennesima struttura - all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sarebbe stato meglio investire del denaro per risolvere tutte le problematiche?

l'attribuzione della qualifica di lavori straordinari per la banda larga, il silenzio assenso nel caso di interventi di questa natura, la velocizzazione delle procedure autorizzative e la riduzione dei termini temporali previsti per le autorizzazioni. È il nostro modo di vedere la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, rispetto al quale, come sapete, come Governo di centrosinistra abbiamo investito risorse ingentissime, miliardi di euro. Adesso è il momento di risolvere i problemi che impediscono lo sviluppo, l'attuazione e l'efficacia di questi provvedimenti che noi avevamo assunto in passato.

difficile comprendere come alcune realtà del territorio possano impedire lo sviluppo complessivo generale dell'Italia. Consideriamo

Non condividiamo, invece, la destrutturazione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Com'è noto, questo Consiglio è formato da esperti che hanno diverse e autorevoli competenze e, senza alcun onere per la finanza pubblica, con i suoi pareri è sempre stato uno strumento di costruzione

con l'approvazione di una nostra proposta abbiamo assicurato la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema emergenza-urgenza, perché abbiamo permesso l'accesso alle procedure concorsuali per la disciplina della medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza al personale medico. Abbiamo garantito questa possibilità. È una buona notizia, sia per la classe medica, che per i pazienti e per tutti coloro che vedono riconosciuto il lavoro egregio e impegnativo che svolgono all'interno del pronto soccorso. Rimane irrisolto il tema della medicina d'urgenza territoriale: il fatto, se pur condivisibile, di aver deciso la possibilità transitoria di assegnare gli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione non risolve tutti i problemi. C'è bisogno anche di altro e, pur apprezzando questo tipo di proposte, aspettiamo che il Governo prosegua nella propria azione, nel confronto che abbiamo avviato Per quanto riguarda, invece, l'articolo 10, non riusciamo a comprendere - ed è uno degli aspetti che hanno reso deforme il provvedimento - che cosa c'entri il reclutamento dei dirigenti scolastici con la modifica della legislazione riguardante il noleggio con conducente: è incomprensibile. Su questo c'è un dibattito nel Paese (abbiamo visto tante proteste anche fuori dall'Aula del Senato) e sono state provocate tante disfunzioni. Noi abbiamo fatto delle proposte per risolvere alcune delle problematiche che ci sono state sottoposte: non sono state accolte, ma le elenco comunque. PRESIDENTE. Senatore

alla propaganda che è stata fatta. C'è poi un emendamento, che è stato presentato in Aula, sullo scorrimento della graduatoria per l'assunzione di agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, un emendamento che modifica le regole di un concorso fatto nel 2017: anche questo è da valutare. Presidente, colgo l'occasione della sua attenzione per sollecitare ancora una valutazione sul fatto che nel decreto-legge siano stati inseriti

che, a nostro modo di vedere, semplificava e sburocratizzava, ciò che avrebbe dovuto essere il senso del provvedimento. Invece questo decreto-legge non solo non raggiunge questo scopo ma, dopo che è stato ingrossato a dismisura, è diventato sostanzialmente un elefante che farà non pochi danni nella delicata cristalliera del nostro Paese. Vi ringrazio per l'attenzione Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

legiferare che non riteniamo opportuno e che non riteniamo garantisca la trasparenza, che invece è il principale scopo dell'esame parlamentare dei provvedimenti.

appalti pubblici, tracciabilità dei rifiuti, edilizia penitenziaria, piattaforme digitali, formazione dei medici, concorsi e formazione dei docenti, e questo solo per toccare i punti principali. Per trovare una forma di omogeneità, e anche per dare un titolo al provvedimento, si è fatto un po' come in quel gioco televisivo, molto carino, dove c'è una serie di parole che sembrano non avere nulla a che fare l'una con l'altra e il concorrente deve trovarne una che invece, per qualche strano ragionamento, possa le altre. Ecco, questo però non è un gioco. Qui stiamo facendo legislazione e siamo particolarmente preoccupati per il fatto che il provvedimento al nostro esame discende da una legge di bilancio, approvata nei modi che sappiamo e che hanno causato i rilievi del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale,

presentare gli stessi provvedimenti con modalità diverse. Non è indispensabile, per la maggior parte di questi, il decreto-legge, perché abbiamo norme di ogni tipo, anche di carattere ordinamentale. Non riteniamo pertanto che questo sia il modo di legiferare per rispetto all'istituzione e per rispetto agli italiani, che hanno il diritto di avere leggi chiare, dove al titolo corrisponda un contenuto e non si ricorra a concetti del tutto astratti e opinabili, come «semplificazione», laddove sappiamo che le leggi di semplificazione tendono a complicare le cose quando poi abbiamo volumi come quello che abbiamo in mano, di 820 pagine, molti dei quali sono stati approvati in Commissione. Non è questo il modo per rendere un servizio al nostro Paese.

autorevole appello, fatto al Governo sul pericolo di una totale spoliazione dei tempi del Parlamento per esaminare quel provvedimento, è rimasto

Oggi temo - mi auguro di no - che si sia alla vigilia di un ulteriore strappo, ma il Senato, per fortuna, Presidente, ha gli antidoti per evitare questo tipo di strappi. Mi riferisco ad una battaglia, che mi sono intestato con il sostegno dei miei colleghi in Commissione, rispetto a un argomento sul quale non abbiamo mai fatto ostruzionismo nel merito, per significare a quest'Assemblea come un decreto-legge di 12 articoli in poche pagine rischi di trasformarsi in qualcosa di diverso, fatto, signor Presidente, da 61 pagine ulteriori e 83 proposte emendative.

al CSM - della configurabilità o no del cambiamento del decreto-legge durante il periodo della sua conversione. Nel 2012 la Corte costituzionale ha

un decreto-legge ha bisogno - come dice l'articolo 77 della Costituzione - di una legge di conversione, quindi che il Parlamento lo trasformi in legge, pena la decadenza,

di un'accelerazione temporale in quanto va esaminato e approvato entro sessanta giorni, necessita di una compatibilità con il testo iniziale del decreto-legge. il decreto-legge si può modificare, ma nella logica della compatibilità e della coerenza o con gli articoli contenuti nel decreto-legge o con le finalità che lo stesso intende portare avanti quando si tratta di decreto-legge *omnibus* come quello attuale, perché è così. Dice la Corte che «Il Parlamento è chiamato a convertire (...) in legge un atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo (...) In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione.

Questo rigore - dice la Corte - era stato ribadito e mai smentito da una delibera della Giunta per il Regolamento del novembre 1984 (Presidenza Cossiga). Per la Corte, quindi, il Senato ha in sé i meccanismi, gli antidoti, la possibilità di decisioni interne per evitare che possa avvenire un'invasione da parte dell'Esecutivo e della maggioranza nei confronti delle regole parlamentari e delle minoranze.

utilizzando un percorso ordinario di conversione in un percorso autonomo per imporre delle regole non discusse nelle Commissioni competenti e non discusse secondo le regole parlamentari. Signor Presidente, noi abbiamo denunciato più volte in Commissione l'anomalia che si stava consumando. Cito alcuni esempi eclatanti: a proposito di prestito all'Alitalia, si introducono norme che modificano la redazione dei bilanci delle banche e delle società finanziarie. All'articolo 5 si parla di semplificazione delle norme sugli appalti pubblici sotto soglia, e si aggiungono articoli aggiuntivi che parlano di patti territoriali, semplificazione in materia edilizia, responsabilità civile in tema di assicurazioni. L'articolo 7 tratta di edilizia penitenziaria? Invece si introducono emendamenti che toccano interventi in zone sismiche, certo interessanti, importanti e urgenti, ma da adottare con un altro provvedimento. L'articolo 8 riguarda piattaforme digitali? No, all'interno si parla anche di semplificazione in materia di cinema e sistemi audiovisivi. L'articolo 9 tratta di formazione specifica in medicina generale, e si aggiungono emendamenti che parlano del carattere scientifico dell'IRCCS, delle farmacie, delle disposizioni anticipate di trattamento, dei LEA.

di una norma che interpreta autenticamente una legge che si occupa di rinnovo degli ordini forensi. Si parla di un emendamento che aggiunge un'unità dirigenziale all'interno del Ministero degli interni per il contrasto all'immigrazione.

ma voglio rivolgermi anche ai colleghi di maggioranza, che hanno insistito pervicacemente, tanto da costringere il sottoscritto a chiedere al Capogruppo di cambiare Commissione, nel dichiarare ammissibili proposte emendative che effettivamente erano

e ritirare alcuni emendamenti per salvaguardare la dignità di questo Senato.

le loro gazzarre nella scorsa legislatura contro l'utilizzo dei decreti-legge da parte del Governo. Sarebbe facile, ma francamente non ne vale la pena. Noto soltanto come cinquestelle e Lega siano riusciti nella difficile impresa di trasformare la loro demagogia di opposizione in una ben più pericolosa demagogia governativa. Ora il punto è un altro. Prescindo dal merito degli emendamenti che in questa fase non rileva, perché qui oggi il punto è che nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento di conversione di un decreto-legge sono state approvate talmente tante disposizioni estranee al suo contenuto da renderlo abbondantemente incostituzionale. Nel febbraio del 2012 il Parlamento è stato formalmente avvisato dalla Corte costituzionale che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché c'è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione. Le Camere possono - lo ha ricordato poco fa il senatore Schifani - certamente emendare i testi dei decreti,

Se il legame di omogeneità tra il decreto e la legge di conversione viene infranto, si realizza per la Corte costituzionale una violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in ragione - e lo cito - di un «uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce». Quelle della Corte sono considerazioni inequivoche, che su questo punto segnano in modo definitivo la sua giurisprudenza. Con la più assoluta chiarezza e con i toni fermi ce l'hanno formalmente ricordato il Presidente della Repubblica, la Giunta del Parlamento e anche, ripetutamente, i Presidenti dei due rami del Parlamento. Il testo approvato in Commissione mostra come per la maggioranza e per il Governo non contino nulla né le sentenze della Corte, né i richiami del Presidente e delle alte cariche istituzionali. non so se sia più grave la violazione della Costituzione o l'arroganza con cui viene commessa: un'arroganza così sfacciata da far pensare alla volontà di ripetere nel futuro analoghe violazioni. Questa mattina un quotidiano riferisce che dai dieci articoli iniziali il testo del provvedimento è arrivato a 61 pagine di emendamenti. un fascio di emendamenti visibilmente incostituzionali per la loro estraneità al contenuto del decreto-legge; ciò nonostante, in Commissione sono stati dichiarati ammissibili e poi approvati dalla maggioranza. Se questi emendamenti saranno approvati anche in Assemblea, verranno macchiate di incostituzionalità parti rilevanti della legge di conversione. Che ci fa nel decreto sulle semplificazioni un emendamento che innalza vistosamente i termini della sanatoria che evita al datore di lavoro le sanzioni per omesso versamento dei contributi? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Che ci fa un emendamento sui bilanci delle banche e delle società finanziarie? Oppure l'emendamento su un posto in più nell'organico del Ministero dell'interno? Il Senato sa bene che le regole per la formazione delle leggi costituiscono un elemento costitutivo degli Stati di diritto. Leggi approvate senza un rigoroso rispetto delle procedure costituzionali sono una caratteristica dei regimi, non delle democrazie. modifiche del Regolamento del Senato approvate nella passata legislatura, c'è la previsione di tempi più ampi per il lavoro delle Commissioni. La modifica ha l'obiettivo di garantire alle Commissioni tutto lo spazio necessario per un esame quanto più approfondito possibile dei provvedimenti, così che possano giungere in Assemblea in una forma ben definita. Più tempo alle Commissioni per migliorare i provvedimenti, non per dare la possibilità a Governo e maggioranza di rimpinzare le leggi di conversione con emendamenti su materie totalmente estranee al contenuto del decreto-legge. Questo è quello che è successo, signora Presidente. Le Commissioni 1a e 8a hanno usato gran parte del tempo loro rimasto dopo il braccio di ferro sulle trivelle per approvare emendamenti incostituzionali. Non viviamo tempi fortunati per il Parlamento. Casaleggio e Grillo prevedono che presto sarà inutile. Il Governo pensa di sostituire la democrazia parlamentare con una democrazia che chiamano diretta e che di democratico non ha nulla. Governo e maggioranza pensano che sia lecito modificare la collocazione internazionale ed europea dell'Italia senza che il Parlamento ne abbia discusso in profondità. E ora la maggioranza sfida la Corte costituzionale approvando una legge di conversione palesemente incostituzionale. Davanti a questa deriva mi sono chiesto chi, qui in Senato, disponga dei poterti necessari per fermarla. Li avrebbero avuti i Presidenti delle Commissioni 1a e 8a, cui spetta il giudizio di ammissibilità degli emendamenti. Ma i due Presidenti hanno rinunciato ad esercitare le loro prerogative. Anche su questo punto ci sarebbe molto da riflettere, considerato come in questa legislatura le Presidenze delle Commissioni stiamo andando sempre più assumendo il profilo di organi dei partiti di maggioranza, così da perdere, parallelamente, il carattere *super partes* proprio del loro ruolo. Signora Presidente, il Regolamento del Senato le affida grandi responsabilità a presidio della qualità dei nostri lavori e, conseguentemente, della costituzionalità delle leggi. pregiudiziale che stiamo discutendo verrà respinta nell'indifferenza della maggioranza. Chiedo, quindi a lei, signor Presidente, di difendere l'onore del Senato e di esercitare tutte le sue prerogative, con quel rigore che è non solo necessario, ma persino obbligatorio, quando risulta evidente che la palese incostituzionalità di vaste parti del provvedimento

a ristabilire alcuni princìpi e alcune regole. Potremmo dire, come si diceva in passato (ritorno allo Statuto): ritorno alla Costituzione.

per cui non solo abbiamo assistito a un abuso della decretazione d'urgenza, ma il punto vero per cui molte volte siamo stati costretti a presentare pregiudiziali di costituzionalità è che tutti i presupposti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione per i decreti-legge nella maggior parte dei casi non erano stati assolutamente rispettati.

che la Corte ritiene implicitamente previsto dall'articolo 77 ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Quest'ultima disposizione, laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo,

di fatto definisce illegittimo *tout court* un decreto-legge che non corrisponde ai requisiti della omogeneità e alla corrispondenza tra il contenuto del decreto-legge e il titolo stesso.

e solo in un caso abbiamo avuto ragione, nel senso che siamo stati ascoltati e la maggioranza ha ritirato alcuni emendamenti che erano tra i più palesemente disomogenei. Pensiamo agli emendamenti sulle donazioni o ad alcune norme di modifica della procedura penale, inserite in una parte riguardante la procedura civile e altro. Ripeto, però, che è stata una piccola parte,

di intervenire, così come prevede il nostro Regolamento. Come organo monocratico ha tutta la possibilità di tentare di riportare la situazione sui binari giusti, ma - torno a ripeterlo

e urgenza e alla mancanza dei presupposti di omogeneità, che la Costituzione prescrive implicitamente, anche nell'articolo 77, e su cui la Corte costituzionale

veramente vedere in quest'Aula questa sorta di mostro, in cui è stato infilato di tutto. Voglio ricordare anche

è stata convocata inutilmente per dare il tempo a questa maggioranza di ritrovare la sua unità momentanea e una quadra. La settimana scorsa - qui ci si dimentica di tutto - noi abbiamo atteso inutilmente questo decreto e poi siamo arrivati a lunedì.

Oggi è stato sottolineato un profilo, con una pregiudiziale di incostituzionalità, e mentre siamo qui a discutere su tale profilo e su tale pregiudiziale, arrivano dei comunicati stampa molto chiari,

infarcito di troppe norme, che arriva in Aula con oltre 80 emendamenti da parte della maggioranza, che quindi continua a emendare se stessa

perché se la quantità di norme non viene ridotta e da questo testo non vengono stralciate alcune di queste numerose norme,

si va dalle norme sulla xylella alle trivelle, dalla *web tax* alle farmacie, dagli NCC alla DURC, passando attraverso IRES, RC auto, etichette dei prodotti alimentari, concessioni autostradali e molto altro ancora. Non vorrei continuare, ma potrei. Vi dovete dare delle priorità

rincorrere sostanzialmente alcune fette di elettorato, peraltro difforme all'interno della maggioranza. Date invece le priorità e le risposte che il Paese richiede.

senatori, nella giornata di sabato, dopo una lunga malattia, è scomparso Giuseppe Zamberletti, parlamentare eletto per sette legislature, più volte Sottosegretario e Ministro della Repubblica. A lui si deve la creazione di una moderna e innovativa Protezione civile. Zamberletti seppe infatti ricavare dalle emergenze progetti e politiche di notevole utilità per l'Italia intera. Ebbe l'obiettivo di ridurre i danni causati al nostro Paese da calamità naturali ed errori e incuria dell'uomo. Lo perseguì con ingegno, competenza e perseveranza ammirevoli. Sin dai terribili terremoti del Friuli e dell'Irpinia, Zamberletti riuscì a mettere a sistema l'attività centrale dello Stato, gli enti locali e il volontariato, attuando quei principi di solidarietà e sussidiarietà che ne hanno sempre ispirato l'impegno politico. Sempre coerente con i suoi valori democratico-cristiani, dedicò tutta la sua attività pubblica al bene comune, con intuizioni che hanno consentito al nostro Paese di essere protagonista nell'azione di soccorso anche nei contesti internazionali. Ai familiari e a tutti coloro che gli sono vicini giungano quindi i sensi del cordoglio e della vicinanza del Senato della Repubblica. Vi invito ad osservare un minuto di silenzio.

questo decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre dell'anno scorso, poi è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e presentato al Senato. Avrebbe dovuto essere un treno ad alta velocità,

altri vagoni, troppi, al punto che il Presidente della Repubblica, da notizie di agenzia, sembra abbia fatto filtrare di non essere d'accordo e di non essere disponibile a firmare un provvedimento che, da decreto di semplificazione, è diventato di complicazione. Quindi, cosa accadrà in queste ore? Accade innanzitutto che stiamo discutendo di un testo e di emendamenti che probabilmente saranno a loro volta ritirati, dopo intese in qualche stanza o bagno di questo Palazzo tra i Gruppi della maggioranza, per evadere un avvertimento significativo della Presidenza della Repubblica. Siete stati colti con le mani nella marmellata.

potrebbe chiamarsi più legittimamente "complicazioni" o "correzioni", perché correggete una serie di provvedimenti che avete fatto male, da quello sulla tassazione per il volontariato al provvedimento sui taxi, dal provvedimento sulla rottamazione alla nuova *web tax*. Avete modificato, pochi giorni dopo la loro approvazione, provvedimenti che voi stessi avete realizzato: una confusione assoluta, in cui voi stessi apparite più che confusi, direi smarriti. Potrebbe chiamarsi anche "decreto *omnibus*", perché nel frattempo avete aggiunto a questo decreto semplificazione la proroga del provvedimento di commissariamento e di finanziamento dell'Alitalia. Che c'entra con la semplificazione? E con quale piano? Senza un piano: proroga e basta, altro denaro pubblico senza dirci in quest'Aula, in sette mesi, cosa volete fare dell'Alitalia. Avete inserito il provvedimento sulle trivelle, che secondo le

che producono, che hanno un'impresa - la cosa peggiore è dire che tra diciotto mesi si cambieranno le norme. È meglio cambiarle subito, perché, se rinviate i cambiamenti di diciotto mesi, nel frattempo si blocca ogni cosa. Lo dico ai parlamentari della Lega: l'associazione degli industriali ha definito questa vostra decisione un suicidio industriale, che permette sostanzialmente alle imprese straniere

su un campo agricolo per impedire che fosse abbattuta una pianta di ulivo che poi ha creato contagio. Il senatore Lello Ciampolillo ha addirittura utilizzato le sue prerogative parlamentari per tutelare quella pianta malata e impedire che fosse tagliata; per questo gli atti sono stati trasmessi alla procura della Repubblica. Con questo provvedimento e non c'entra nulla - voi prevedete un nuovo reato, punito con il carcere da uno a cinque anni, per chi non abbattere gli ulivi colpiti dalla Xylella.

"decreto figuraccia", perché tra poche ore dovrete cambiarlo di fronte al richiamo del Capo dello Stato. Voi giocate con le parole, come avete fatto nel caso del decreto dignità,

cento. Effetto del decreto dignità? Forse. Effetto dell'annuncio del reddito di cittadinanza, perché ciascuno si sta collocando in una posizione tale per poi ottenere il reddito di cittadinanza? Forse. Voi avete creato un pasticcio parlamentare e una confusione legislativa tali per cui ora ne pagherete le conseguenze, con la figuraccia che farete nelle prossime ore per ritirare gli emendamenti che avete già presentato e per snellire questo provvedimento. Credo che questo sia l'esempio più classico di quanto non avreste dovuto fare, mentre per confusioni interne siete entrati nella paranoia elettorale per cui ciascuno insegue l'altro - avete consentito al Parlamento di creare questo obbrobrio. Noi non lo permetteremo più.

quello che stiamo per approvare è un provvedimento importante e strutturato. Il Parlamento è chiamato a trasformare in legge un decreto-legge di cui il Paese ha effettivamente bisogno. Parliamo di misure per il sostegno e la semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, vale a dire un provvedimento di cui abbiamo bisogno come l'aria da respirare dopo dieci anni di crisi finanziaria e, soprattutto, dopo sette di Governo PD. La volontà del nostro Governo, sottoposta al giudizio del Parlamento, è quella di intervenire su alcuni specifici settori che oggi si ritrovano a dover operare in oggettive difficoltà normative. Il decreto-legge semplificazioni vuole andare incontro alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in vari campi: dalle agevolazioni economiche per l'accesso al credito alle semplificazioni procedurali per la gestione dei rifiuti, dalle regole per la partecipazione agli appalti pubblici all'accessibilità delle piattaforme digitali ministeriali, dalla semplificazione del campo delle assunzioni nel mondo della sanità e dell'istruzione ad una migliore normativa per gestire l'edilizia penitenziaria sia quella esistente, che quella necessariamente programmata. I passaggi istituzionali che abbiamo compiuto fino ad oggi qui in Senato per la conversione di questo decreto-legge si sono svolti in un clima di correttezza di cui, per onestà intellettuale, devo dare testimonianza per quanto riguarda il rapporto tra maggioranza e opposizione.

Ne è uscito un testo a nostro avviso migliore, maggiormente completo, che sviluppa i dodici articoli di cui è composto in modo armonico, integrandoli in alcune parti e fornendo quelle risposte ai problemi che, come sistematicamente accadeva con la sinistra al Governo, venivano lasciati in una sorta di limbo, senza essere risolti o nemmeno affrontati perché probabilmente ritenuti troppo complessi. Un esempio lampante è quello del blocco delle assunzioni delle forze dell'ordine, follia che ha generato uno squilibrio che stiamo quotidianamente scontando e che ci ha costretti ad agire con tempestività per andare a ristabilire un livello occupazionale minimo in grado di sostenere l'intero settore. Questa emergenza, iniziata con i Governi di sinistra per i quali la sicurezza evidentemente era un qualcosa che aveva importanza relativa, ci ha quindi obbligati ad una precisa scelta: fare un nuovo concorso, rimanendo ancora fermi ad aspettare tempi lunghi e incerti, oppure andare ad assumere nuovi agenti fin da subito, attingendo dalle graduatorie esistenti, rispettando però le regole vigenti e dunque quelle limitazioni in termini di età e titoli di studio, secondo le modifiche introdotte escludendo di fatto una parte delle persone che avevano partecipato all'ultimo concorso senza ovviamente risultarne vincitrici. Ancora una volta, quindi, ci siamo trovati a dover gestire problemi causati dai Governi precedenti, cercando la soluzione migliore per il Paese. però il fatto che se si fossero fatte le assunzioni per tempo non sarebbe sorto nemmeno il problema e il Partito Democratico avrebbe potuto cambiare la legge - come effettivamente ha fatto - senza escludere centinaia di persone dalla graduatoria. Si promettevano nuovi agenti ma, alla fine, non si assumevano mai perché - veniva sempre risposto - mancavano i soldi. Già, mancavano sempre i soldi per assumere agenti; l'Europa chiedeva rigore nei conti, ma si poteva però chiedere flessibilità per dare gli 80 euro, vero? c'è una novità: noi siamo differenti, noi gli agenti li assumiamo sul serio. In questo provvedimento c'è molto altro ancora e faccio alcuni esempi. Sugli enti locali, per esempio, andremo a fornire ulteriore ossigeno ai Comuni, ripristinando completamente il fondo IMU-TASI che il Governo precedente aveva deciso di interrompere a fine 2018, ma che noi, ritenendolo di importanza basilare, già avevamo parzialmente finanziato per il 2019 nella legge di bilancio a fine dicembre.

Fatti, non promesse, che certificano il nostro sostegno agli enti locali, troppo spesso dimenticati (per non dire proprio massacrati) dai vari governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni Nella trasformazione in legge di questo decreto-legge, vorremmo (e vogliamo) andare a far seguire i fatti alle parole per quanto riguarda i superstiti ed i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano, andando a stabilire indicazioni semplici per i risarcimenti dovuti. È nostra intenzione fornire risposte semplificative anche per quanto riguarda il tema dell'etichettatura alimentare, in quanto riteniamo che sia un sacrosanto diritto dei cittadini avere informazioni semplici e veritiere in merito a ciò che finisce sulle loro tavole. È di tutta evidenza, quindi, che trasformando in legge questo decreto-legge vogliamo apporre alcune significative ed importanti migliorie, ma non si possono elencare tutte nei pochi minuti a disposizione. Dobbiamo però citare ancora il ripristino dell'IRES agevolata per le associazioni *no profit* e la nuova normativa per gli NCC, la semplificazione introdotta per gli ordini degli avvocati, il passaggio della gestione delle concessioni idroelettriche alle Regioni (avanti verso l'autonomia regionale).

per un reale sostegno ed una effettiva semplificazione cui prestissimo dovranno seguire altre misure che, mi auguro, potranno partire proprio dal Parlamento già dalle prossime settimane perché, come Lega, abbiamo in mente diversi interventi che, ne siamo certi, gli italiani aspettano da almeno sette anni.

nell'affrontare questa discussione penso sia oggi difficile parlare di semplificazione perché il provvedimento in esame contiene molte cose, troppe. ormai un provvedimento *omnibus* e di semplificazione c'è poco o niente. Vedete, quando si parla di semplificazione si immagina che si proceda nel cancellare norme e leggi che opprimono la vita di cittadini e aziende, una burocrazia con più di 110.000 leggi fra cui ancora centinaia di quando questo Paese era governato da un re. Invece di semplificare, discutiamo un provvedimento che è un vero e proprio pentolone di norme eterogenee ma che ha un nome accattivante: «semplificazione». Nella pratica non c'è minimamente l'intento di snellire norme che appesantiscono le operazioni della pubblica amministrazione, una strategia comunicativa che, come in altri casi, si concentra su un messaggio semplice ma efficace intorno a provvedimenti con poca sostanza o spesso con norme non pertinenti. Una scena già vista: decreto sicurezza con poca sicurezza, decreto Genova con poca Genova, decreto dignità con poca dignità, così un decreto semplificazione con poca semplificazione. Grandi titoli, pochi contenuti. Come sempre, la disorganizzazione nel programmare i lavori nelle Commissioni, poi, regna sovrana e i contrasti interni alla maggioranza hanno tenuto in ostaggio quest'Assemblea per giorni: sospensioni e rinvii continui. Più che un decreto semplificazione, un decreto confusione. Così come si ripete la scena di una maggioranza le cui forze litigano tra di loro, che presenta tutta una serie di emendamenti fra i più variegati che poco c'entrano con la semplificazione: penso alla moratoria ai permessi di ricerca ed estrazione di gas e petrolio; penso all'emendamento riguardante le imprese che si occupano di economia circolare,

Non dimentichiamo poi l'emendamento sul taglio dell'IRES che avete dovuto presentare per rimediare al grossolano errore fatto sempre da voi nella legge di bilancio, dove avete penalizzato il volontariato.

Un caos normativo, quindi, su un provvedimento che teoricamente dovrebbe avere il fine ultimo di snellire le procedure. Infine, vi sono gli emendamenti che riguardano la Xylella e le gelate in Puglia un intervento corretto ma tardivo per tamponare il disinteresse di una legge di bilancio in cui l'agricoltura è stata completamente dimenticata, oppure quello che chiede l'etichettatura con l'indicazione di origine italiana dei prodotti usati nelle lavorazioni, sicuramente positivo e condivisibile, ma parziale. Colleghi, l'agricoltura, insieme alla pesca e all'agroalimentare italiano, hanno bisogno di una vera e propria opera di semplificazione. Occorre un'analisi che possa portare alla cancellazione di norme, leggi e atti burocratici che soffocano l'attività di migliaia di piccoli e medi agricoltori e pescatori. Norme che spesso alimentano la burocrazia e impediscono la vera attività produttiva. Questo significa semplificare: alleggerire l'attività di chi produce ricchezza per la nostra Nazione. Oggi, fuori di qui, i nostri agricoltori e i nostri pescatori vivono una realtà in cui far sopravvivere le proprie aziende è sempre più difficile. Non hanno bisogno di illusioni semplificative; hanno bisogno di concretezza, di quella concretezza che sempre caratterizza chi con la terra e il mare lavora ogni giorno. Ma tutto questo avrebbe bisogno di approfondimenti nelle competenti Commissioni per riuscire a varare norme veramente condivise ed efficaci per il settore. Quello che non è più accettabile è questa continua azione di cui non si intravede un progetto compiuto per il sistema paese: un'azione politica che sembra piuttosto finalizzata a una strategia puramente elettorale, fatta di *spot*, per accontentare portatori di interessi e ottenere consenso. In conclusione, Presidente, l'agricoltura, la pesca e la caccia hanno bisogno di una strategia complessiva e non di interventi *spot*, con emendamenti solitari a qualche provvedimento di carattere generale. In questa maniera si possono mettere solo delle toppe, che, come tutte le toppe, lasciano il tempo che trovano. Non abbiamo bisogno di toppe, ma di una pianificazione complessiva e strategica che guardi in maniera compiuta al futuro di questi comparti, e in generale della Nazione. La politica delle toppe non è la politica di Fratelli d'Italia. Non è la politica che serve alla nostra Nazione.

«La casa è mia. Provate a toccarla… Fa' tanto di avvicinarti e t'ammazzo come un cane. Ma non son io, io non posso far niente, io perdo il posto se non eseguo gli ordini. Del resto, cosa credete di risolvere ammazzando me? Vi impiccheranno, certo, ma prima ancora d'impiccarvi ne manderanno un altro qui, con la trattrice, a buttarvi giù la casa. Come vedete, è inutile ammazzare me. "Vedo", chi te li dà? Vuol dire che andrò a scovare lui. È lui che ammazzo". Non volete proprio capire: anche lui riceve gli ordini dalla banca. La banca dice: sbatti fuori quella gente, abbatti la casa o ci rimetti il posto. Ma ci sarà pure un presidente, una direzione; io prendo il fucile e vado alla banca a fare una carneficina. Ma anche la banca, da quello che so, riceve gli ordini… Gli ordini dicono: o ci mostrate gli utili, o vi mettiamo in liquidazione. Ma da chi si deve andare allora, maledizione? Ci sarà pure un responsabile da far fuori. Io non ho nessuna intenzione di crepare di fame senza ammazzare chi mi assassina. Non so cosa dirvi. Forse non esiste un responsabile da poter far fuori… Probabile che, come dite responsabile di tutto è la proprietà.». Cari colleghi, sicuramente avrete tutti intercettato questa pagina tratta da «Furore» di Steinbeck, un grandissimo romanzo che avvitava nella letteratura il racconto della grande depressione americana (era il 1939). Io quella pagina l'ho recuperata tante volte. Una delle ultime volte è stata quando

è dalla storia di Sergio Bramini che nasce anche un impegno politico per modificare l'articolo 560 del codice di procedura civile. Sergio ormai è diventato un emblema. Qualcuno diceva: «vi fate la passerella davanti alla casa di Sergio Bramini». Come vedete, il fatto che noi oggi cambiamo quell'articolo 560 significa che non abbiamo fatto alcuna passerella: vuol dire che Di Maio e Salvini, quando andarono a trovare, con me e con altri, Sergio Bramini, volevano incidere profondamente

la corda che lo hanno impiccato. E lui, pur di non mandare a casa i dipendenti - perché gli imprenditori veri rispettano i propri dipendenti, perché gli imprenditori veri di questo Paese conoscono vita, morte e miracoli dei loro lavoratori e dipendenti - cosa ha fatto? Ha impegnato la propria abitazione. Questo forse nel Paese che ci state consegnando, è un peccato mortale, perché poi effettivamente Sergio è stato sloggiato, scaraventato fuori a seguito di una norma che io considero ingiusta, e per questo mi sto impegnando con voi, con la maggioranza, a cambiarla. Quello che accade è il frutto è il frutto di una intossicazione neoliberista; è il frutto di un racconto malato, di un racconto per cui le sofferenze bancarie sono diventate più importanti di coloro che soffrono. Colleghi, questo mi fa uscire matto! Le sofferenze bancarie diventano centrali nel racconto della politica, nelle attenzioni della politica, e questo fa scomparire colui che soffre. Guardate che non stiamo anestetizzando l'ipoteca e i suoi effetti: vogliamo soltanto riequilibrare; vogliamo soltanto il buon senso; vogliamo che ciò quando e se deve accadere - soltanto dopo la vendita dell'immobile. Non capisco il motivo per cui bisogna accanirsi e sloggiare, cioè buttare fuori di casa, delle persone quando ancora l'immobile non è stato venduto all'asta. Questo è ingiusto ed è questo il tema: le sofferenze non posso venire prima altrimenti accade che, oltre alle oltre alle sofferenze e ai sofferenti, si genera una insofferenza che diventa insofferenza insofferenza sociale, ed è quella che scatena una battaglia tra l'ultimo e il penultimo. Dentro quelle sofferenze e dentro quei sofferenti c'è un pezzo di classe media del Paese che sta scivolando sempre più nella povertà. Ma io non posso scaraventare fuori di casa e sloggiare le persone quando ancora l'immobile non è venduto, altrimenti dobbiamo fare i conti con delle storie tragiche di gente che è costretta addirittura a dormire in macchina. Qual è allora la dignità? Qual è la crisi che può permettersi di cancellare la dignità delle persone? Noi non lo possiamo accettare! M5S)*. Il racconto di questi mesi e di questi anni ci ha consegnato fondi locusta, fondi avvoltoi. Il bestiario finanziario è un bestiario che che ammalora, che aggrava ancora di più la sofferenza di persone che, come nel caso di Sergio, si sono ritrovate a dover fallire per colpa di uno Stato che non pagava. Oggi per fortuna, grazie a questo Governo e a questa maggioranza, finalmente i debiti della pubblica amministrazione verranno pagati *(Applausi dal messi a disposizione di questi imprenditori, ma ci sono anche famiglie che, per colpa della crisi, non sono riuscite a fare fronte ad un impegno con le banche.

perché non c'è più posto». In questa maggioranza noi siamo, con questo Governo, l'ABS sociale.

il decreto-legge «semplificazione», come i decreti-legge «dignità», «sicurezza», «spazzacorrotti» o «concretezza», ha nel titolo una buona comunicazione: genera aspettative che diventano illusioni, ma nel frattempo queste illusioni lasciano l'Italia più sola e le persone più fragili; lasciano le famiglie e le imprese meno sicure nell'affrontare il loro futuro. Quando la comunicazione verrà finalmente sostituita dalla rendicontazione, cadranno utopie e illusioni che nel frattempo avete generato. La realtà mostrerà, purtroppo per l'Italia, il suo volto. Onorevoli senatori, come già è evidente, aumentano le domande di disoccupazione. Veniamo via via spinti verso una nuova recessione e il decreto semplificazione si trasformerà in nuove complicazioni per famiglie ed imprese, anche perché è stato riempito in maniera assurda, a volte anche abnorme e in contrapposizione con l'entità stessa del da innumerevoli iniziative legislative. Ne parleremo più approfonditamente nella discussione in merito agli emendamenti. Abbiamo apprezzato la proposta del presidente Patuanelli di eliminare dal decreto semplificazione la questione riguardante la modifica del codice degli appalti. Tuttavia, riteniamo che siano tante le materie che sono state introdotte, a cominciare da quelle più delicate e pertinenti per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese: mi riferisco alle grandi questioni energetiche che avete deciso di affrontare nel provvedimento. Insomma, l'Italia richiede una politica energetica nazionale ed è proprio nella riconversione in chiave ecologica dell'economia che si genererà nuova occupazione e nuovo sviluppo. Questo avrebbe richiesto una misura organica e non misure, come quelle contenute nel decreto semplificazione, finalizzate ad aprire conflitti più che a risolvere problemi: conflitti tra lo Stato e il mercato o tra il pubblico e il privato, tendenti tutti,

Tante sarebbero state le misure che avrebbero richiesto provvedimenti organici e che questa la maggioranza ha deciso di introdurre impropriamente all'interno del decreto. Penso sia importante una semplificazione degli emendamenti per ripristinare, anche costituzionalmente, la coerenza necessaria tra un decreto-legge approvato molti mesi fa mesi fa e l'atto parlamentare che si sta discutendo in fase di conversione. Serve un riallineamento che mi auguro troverete nelle prossime ore.

anche in relazione a tanti emendamenti che in quella sede e in quella fase non furono accolti; con superficialità e continuando da parte della maggioranza un'opposizione al passato non sono stati recepiti fin dalla legge di bilancio. Mi riferisco a due questioni fondamentali: IRES ed enti locali. Nel caso dell'IRES emerge, a mio avviso, un dato oggettivo: abbiamo sostenuto da sempre che la povertà non si sconfigge per decreto; che la solitudine e le fragilità richiedono un lavoro, non i sussidi; che le povertà hanno come denominatore comune una questione culturale e dunque necessitano di formazione. Serve la presa a carico delle persone sole e fragili e dunque serve una dimensione territoriale della presa a carico. Non bastano i centri per l'impiego e le riforme, pur necessarie, che dovranno interessarli; serve un'alleanza tra il pubblico, il volontariato, il *no profit*. Voi, con la legge di bilancio, volevate raddoppiare le tasse alle associazioni che nei nostri territori contribuiscono ad alleviare la solitudine, a contrastarla e a generare accoglienza e presa in carico. Noi, con il nostro emendamento, che oggi avete sostenuto e condiviso, ripristiniamo, a mio avviso con correttezza, una giusta alleanza tra lo Stato, le istituzioni, la società e la comunità. Quella era una tassa ingiusta, che in questa sede deve essere cancellata e che l'iniziativa del Partito Democratico ha contribuito a cancellare.

che oggi sono state recepite all'interno di questo provvedimento. Mi riferisco alla scelta di allora, a mio avviso sbagliata, di non dimensionare correttamente il ristoro del fondo IMU-TASI. Non è vero che c'era una responsabilità dei precedenti Governi: è stata la legge di bilancio ad introdurre una diminuzione di quel fondo; oggi, grazie a una proposta emendativa accolta all'interno di questo provvedimento, ripristinate correttamente una detrazione per gli enti territoriali. Le due questioni che ho affrontato (IRES ed enti territoriali) mostrano una necessità: non c'è una scorciatoia per generare accoglienza e contrastare solitudine e indifferenza; occorre ripartire dal territorio e farlo insieme, in un'alleanza tra Stato, associazioni ed enti locali.

a mio avviso troppo rapida - a dimostrazione che, se si ascoltano anche le proposte dell'opposizione, si possono migliorare i provvedimenti legislativi e non necessariamente si deve continuare a operare in un'opposizione che guarda al passato e non al presente e al futuro di questo Paese.

Signor Presidente, gentili colleghi, sta per finire gennaio e questo provvedimento, insieme a quelli che arriveranno nelle prossime settimane, segna una discontinuità netta rispetto al passato e rispetto a una consuetudine negativa, cui purtroppo sembrava non si potesse trovare una cura. Questo per anni è stato il periodo in cui i partiti tradizionali "davano il La" al "*festival* dei favori" per agevolare questo o quell'amico. So che molti dei miei colleghi che sono stati in maggioranza negli ultimi anni se ne dispiaceranno, ma tant'è. Dovrete abituarvi all'idea che al centro dell'azione politica del Parlamento ci deve essere il cittadino e l'interesse generale; certamente non i particolarismi. Questa aberrazione di inizio anno, come è chiaro, non avverrà quest'anno perché nel decreto-legge semplificazione si interviene invece opportunamente a chiarire e a modificare norme che da anni bloccano vari ambiti della pubblica amministrazione, con interventi mirati che daranno risultati tangibili già nel breve periodo. Questo provvedimento è un aiuto a chi è in difficoltà, spesso non per colpe proprie. Tutte le piccole e medie imprese che hanno dei crediti verso la pubblica amministrazione saranno tutelate da un fondo creato *ad hoc*, che supporterà tante realtà imprenditoriali del nostro Paese nella restituzione dei loro debiti verso le banche. In chi siede tutt'ora in Parlamento e ha assistito negli anni, senza far nulla, a notizie di decine e decine di imprenditori falliti per colpa dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione oggi dovrebbe scattare quantomeno un sentimento di profonda vergogna, veramente profonda. Ne approfitto per un ringraziamento al collega Paragone, che tanto si sta spendendo su questo argomento e sul quale, sono sicuro, non indietreggerà neanche di un centimetro, né oggi, né in futuro. Non solo le piccole e medie imprese: il Governo e la maggioranza si sono già dimostrati attenti e scrupolosi nell'intervenire puntualmente in presenza di tragedie e calamità naturali. È un fatto la pianificazione e l'attuazione in pochi mesi di un piano strategico per la ricostruzione del ponte di Genova. Purtroppo, però, ci siamo trovati ad affrontare e gestire il futuro di chi è stato colpito negli anni passati da eventi calamitosi e non ha ricevuto nulla dallo Stato. Chi ha governato il Paese negli ultimi anni non ha voluto tendere una mano a chi si è trovato vittima di eventi che esulano totalmente dalla propria volontà; per questo è bene ribadire che queste persone devono necessariamente essere supportate da un Parlamento e da un Esecutivo che non possono fare sempre e solo il minimo indispensabile e limitarsi al cordoglio. In questo provvedimento inseriamo, perciò, un aiuto per quelle famiglie che sono state devastate dalla valanga del gennaio 2017 a Rigopiano; si tratta di un gesto che arriva dopo i provvedimenti inseriti nella legge di bilancio, con la proroga della zona franca urbana, indispensabile per tutto il cratere appenninico, nonché la proroga delle assunzioni straordinarie, della sospensione del pagamento dell'IMU e dei mutui per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia del 2012. Il testo oggi in discussione è la prosecuzione naturale di un lavoro che stiamo portando avanti da mesi da mesi e in esso siamo coerenti con la nostra storia e con le battaglie che da sempre il Movimento porta avanti. Finalmente si pone un freno a tutte le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio nazionale, attività che non rivestono carattere strategico per il nostro futuro. Il perché di tutto ciò va ricercato nella politica confusionaria, senza un piano strategico, che gli scorsi Governi hanno attuato nel rilasciare le autorizzazioni per le trivellazioni; un piano, invece, che questo Esecutivo ha perfettamente chiaro e punta alle fonti rinnovabili, in antitesi rispetto al recente passato. una idea di Paese che punta decisa alla decarbonizzazione e al superamento di tutte le fonti energetiche fossili, in una transizione organizzata e condivisa tra Governo ed enti locali. Fino a che non verrà definito il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, tutte le autorizzazioni già rilasciate verranno sospese, insieme ovviamente a tutte le richieste per nuove prospezioni. Sono sinceramente curioso di capire cosa si inventerà domani un certo tipo di stampa per travisare la chiarezza di questa norma; chiarezza che è la stessa espressa dal ministro Costa sull'argomento e che non lasceremo solo in questa battaglia. Già nel mese di ottobre il ministro Di Maio è riuscito a bloccare le trivellazioni in Provincia di Modena e Reggio Emilia, sulle quali ho sottoscritto una interrogazione parlamentare insieme alla senatrice Mantovani, e con il provvedimento in esame blocchiamo decine di richieste di ulteriori autorizzazioni. La voce dei cittadini che da anni ci chiedono di fermare questo scempio del nostro territorio finalmente verrà ascoltata. Nessuno fingerà più che le trivellazioni siano strategiche per la crescita nazionale; nessuno subordinerà più il rispetto dei territori alla volontà di un Ministero in passato governato da poteri esterni alla politica. Il 2019 non poteva iniziare in maniera migliore per tanti italiani: lotta alla burocrazia, protezione verso il territorio e, nelle prossime settimane, la lotta contro la povertà con l'arrivo del reddito di cittadinanza: un aiuto per tanti cittadini che viene invocato da anni

Sono i controlli che faranno la differenza, con pene severe per chi cercherà degli stratagemmi per ottenere il non dovuto. Il fatto che qualcuno tenterà di non comportarsi bene non deve farci restare immobili senza pensare a milioni di cittadini che davvero faticano. Il primo cambiamento deve passare da noi stessi: tutti noi siamo la società ed una società giusta vede i propri componenti rispettarne le leggi. Nel caso si fosse giustamente sanzionati per qualche infrazione, si deve procedere al pagamento senza domandarsi se in quel tal ufficio ci possa essere qualcuno che ci favorisca. I furbi non devono trovare chi li asseconda: questo principio è di una semplicità disarmante. Invito chi si straccia le vesti di fronte a queste norme di buon senso che aiutano tanti italiani a rileggere i dati dell'Oxfam di pochi giorni fa. Vorrei sapere se per voi è un Paese giusto quello che vede il 5 per cento della popolazione possedere la ricchezza di quasi il restante 95 per cento. Lo ripeto: vorrei sapere se per voi è un Paese giusto quello che vede il 5 per cento della popolazione possedere la ricchezza di quasi il restante 95 Vorrei sapere chi ha il coraggio di essere contento di una situazione così allarmante. Spero per questo che si torni tutti a ragionare sul significato delle politiche pubbliche, politiche che devono necessariamente tendere al benessere della più larga parte di popolazione possibile.

strizzare l'occhio all'uno o all'altro secondo le convenienze delle forze della maggioranza. C'è però un tema su cui davvero esame semplifica il lavoro: semplifica il lavoro delle mafie. Lo voglio dire con grande chiarezza e non facendo una battuta, e cercherò di dimostrarlo.

per consentire loro di velocizzare quegli appalti; nulla di tutto questo è stato fatto. Si è fatto dunque un regalo, non c'è traccia delle cose che avevate detto sarebbero state introdotte, e viene confermato che al di sotto dei 150.000 euro gli appalti

di legge spazzacorrotti, ma oggi create le condizioni per aumentare la discrezionalità e diminuire la trasparenza nell'affidamento degli appalti.

che punisce il voto di scambio, ovvero voti in cambio di favori. Avete voluto dimostrare che su questo bisogna fare "il più uno" e ora consentite, con la norma citata, di sgombrare la strada a chi, in cambio di voti, potrà ottenere appalti. Gran parte degli scioglimenti dei Consigli comunali sono avvenuti per questo, perché, con gli affidamenti diretti, i sindaci, in cambio di voti, consentivano alle mafie e ai corrotti di avere quello che volevano. Ebbene, questo è il punto, ma non c'è solo questo.

quello che tratta i temi della sanità, sempre che non rientri nei 40 emendamenti che voi vi accingete a cassare, nel qual caso avremo fatto un minimo di esercizio dialettico.

dove autorevoli fonti parlano della mancanza di circa 15.000 medici per effetto di una sorta una sorta di tempesta perfetta che mette insieme numerose cause, tutte comunque che contribuiscono a creare un potenziale gigantesco pericolo per il nostro Servizio sanitario nazionale, che proprio quest'anno celebra i suoi quarant'anni, tra pregi e difetti.

per rimanere in termini medico-sanitari - da curare sintomi ma non la causa, il malessere di fondo. Viene aperta all'esercizio della professione medica una sorta di *deregulation* che risponde certamente, a modo suo, a l'esigenza reale di garantire i numeri

un infarto: è evidente il bisogno di avere più medici dell'emergenza-urgenza e certamente aprire questa professione a medici non specializzati nell'emergenza è una è una vicenda che crea non poche perplessità, anzi desta una sincera preoccupazione. Oltretutto, tutta questa partita è gravata da una una malinterpretazione: il problema della disponibilità di specializzati fa riferimento alla necessità di ampliare i numeri delle scuole di specializzazione. Aprire una materia così delicata a persone non specializzate dovrebbe, quantomeno, imporre l'obbligo che esse ottengano una specializzazione. Sarebbe anche possibile fare ciò a costo zero, visto che quelle persone, comunque, sarebbero pagate dal Servizio sanitario nazionale e dovrebbero essere obbligatoriamente inserite, magari in soprannumero, nei corsi di specializzazione specifica, ma questo passaggio non è previsto. Questa non è, colleghi,

Io spero che questo sia solo un primo passo, nel senso che si cura con l'aspirina una grave malattia in attesa di individuare, magari, terapia antibiotica giusta - uso sempre termini utili allo scopo - ma questo non c'è nel testo. Non c'è una promessa di provvedere con un provvedimento di sistema a colmare le lacune dei medici, a spazzare via la follia del numero chiuso, aprendo magari

è in grado di far saltare il Sistema sanitario nazionale.

difficoltoso lavoro che le Commissioni hanno svolto, per il quale voglio ringraziare i due presidenti Coltorti e Borghesi e anche la relatrice Pirovano, che hanno consentito di accogliere le istanze

che guarda non soltanto alla fondatezza della decretazione d'urgenza, ma anche alla coerenza nello sviluppo del lavoro parlamentare rispetto al decreto-legge partorito dal Governo, invito le opposizioni a fare chiarezza al loro interno. Infatti, se prima presentano un numero consistente di emendamenti, poi non possono proporre una questione pregiudiziale, anche perché il decreto-legge si sta

abbiamo parlato anche della possibilità di utilizzare e sfruttare un'occasione che madre natura può darci in Italia e non possiamo assolutamente sciupare. Diciamo sì a questa fase di transizione, ma in maniera razionale, con buonsenso e senza mettere in difficoltà tanto i nostri industriali quanto i nostri lavoratori. Mi perdonerete non possiamo farlo - da parte di chi ha fatto trivellare il nostro Paese in mare e in terraferma calpestando tanto la salute dei cittadini quanto l'ambiente dei nostri territori. tratta di un equilibrio che è stato raggiunto tra due forze di maggioranza, due forze politiche che hanno messo al centro buon senso, senso di responsabilità, ma anche coerenza. Un altro aspetto che sfugge in questo dibattito, è che il decreto semplificazioni è coerente rispetto a quanto fin qui il Governo e la maggioranza hanno fatto: si cerca di ridurre la burocrazia e le spese e si cerca di sostenere soprattutto i più piccoli o, meglio, chi è in sofferenza e in difficoltà. una serie di provvedimenti che sono stati varati con la finanziaria. Ma, quando con il decreto semplificazioni si tende una mano alle piccole e medie imprese vittima dell'inefficienza della pubblica amministrazione, le quali per andare avanti e pagare gli stipendi hanno dovuto contrarre un mutuo, questo è un punto di buon senso; è un punto di coerenza rispetto ai provvedimenti che fin qui abbiamo adottato, che richiede sicuramente la decretazione d'urgenza. Quando si mette mano al mercato del lavoro e si toglie un altro pezzo del Jobs Act, che tanta sfortuna ha dato all'Italia e ai lavoratori italiani; quando si elimina il libro unico del lavoro, perché inutile e costoso, questo è un passaggio di buon senso; ed è un passaggio di buon senso anche coerente, perché va nella direzione del decreto dignità. Solo chi è in malafede non può vedere i numeri che il Veneto ha registrato, dimostrando che sono aumentati di gran lunga

Spesso per tanto tempo, per troppo tempo, la burocrazia, e quindi l'appesantimento dei vari gangli del potere, e la precarietà sono state fonti di consenso elettorale. Quell'epoca ora è terminata, perché vogliamo sostituire

si cerca di accelerare la costruzione di nuove carceri e di fare manutenzione straordinaria su quelle esistenti, dando competenze dirette al Ministero della giustizia, in modo particolare al DAP. Merita decretazione d'urgenza un provvedimento che guarda alla dignità, perché combatte il sovraffollamento carcerario, dando appunto dignità tanto ai carcerati, quanto alla Polizia penitenziaria che lavora in queste carceri? C'è poi un'altra questione, la riduzione delle soglie per gli affidamenti diretti. Io ritengo che la posizione presa dalle opposizioni sia assolutamente abnorme, illogica e non coerente con la realtà,

non per fare gli sporchi interessi di qualche malvivente, ma per mettere in circolo economia e moneta per aiutare le imprese e offrire servizi ai propri cittadini. Evidentemente qualcuno è animato da malafede, ma non è così, anche perché la malavita (la criminalità organizzata e non solo) ha fatto le sue migliori fortune anche quando queste soglie erano di gran lunga più basse. È giusto che diciamo di cosa parliamo, però. Con 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto

tra almeno dieci ditte. Vogliamo bloccare l'economia perché ci sono paure, pretesti o pregiudizi? Noi vogliamo far prevalere il coraggio. *(Applausi dai facendo delle regole che imbrigliano l'azione politica nella burocrazia. Si combatte la malavita, così come abbiamo voluto fare con lo "spazza corrotti",

le attuali opposizioni non si sono disarmate del libro dei sogni che hanno dispensato agli italiani, sia quando erano al Governo, sia oggi che sono all'opposizione.

Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il decreto-legge che stiamo esaminando prevede una serie di interventi mirati alla semplificazione e al sostegno di importanti settori della vita dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni; un provvedimento che mostra, nella generalità della sua struttura, il decisivo cambio di passo e di velocità che il Governo e la maggioranza intendono sostenere per favorire la crescita della nostra società. Voglio soffermarmi anch'io, in particolare, sull'importanza della disposizione normativa introdotta dall'articolo 1, per gli effetti positivi e tangibili che avrà sulla vita di tantissime persone, e soprattutto su quella parte sana e produttiva del Paese,

tutte le piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni che, a causa dei ritardi nei pagamenti dei crediti da esse vantati, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti precedentemente contratti con banche o intermediari finanziari vigilati. La sezione speciale del Fondo interviene rilasciando una garanzia al soggetto (banca o intermediario finanziario) che ha erogato il prestito che l'impresa ha difficoltà a restituire. Si tratta, in sostanza, di un sostegno pubblico accessibile alle imprese che dimostrano l'esistenza di un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la difficoltà o impossibilità di restituzione di un precedente finanziamento. un intervento assolutamente necessario in tempi in cui la vita dell'imprenditore è una sfida continua. Chi oggi mette su un'azienda sa bene che cosa significano la fatica, la passione, i sacrifici. Si è costantemente messi alla prova da situazioni complicate, che portano paure e preoccupazioni. C'è la paura di non riuscire ad arrivare ad un fatturato soddisfacente o di non riuscire a recuperare in tempo i propri crediti per rispettare le strette scadenze delle rate di finanziamenti contratti per poter mantenere l'attività, la propria famiglia e la famiglia dei propri dipendenti: la paura, insomma, di fallire, di perdere qualcosa o addirittura di perdere tutto. Per decenni la cronaca ci ha raccontato storie scandalose di imprenditori disperati costretti a prendere atto del fallimento del proprio lavoro, della propria impresa intesa come progetto che tiene insieme reddito e senso di vita. storie di cittadini che rappresentano la vita imprenditoriale del nostro Paese, abbandonati a se stessi da una politica che per troppo tempo è rimasta sorda alle richieste di sostegno e al rispetto delle regole. Tutti conosciamo la triste storia di Sergio Bramini, imprenditore fallito e sfrattato da casa, nonostante vantasse crediti nei confronti dello Stato per oltre 4 milioni di euro. Il MoVimento 5 Stelle e il ministro Di Maio hanno fortemente voluto la nomina di Bramini, che rappresenta il simbolo degli eroi italiani che si battono ogni giorno per la sopravvivenza della propria attività, come consulente del Ministero dello sviluppo economico per lanciare subito un messaggio di speranza, ma soprattutto per trovare soluzioni concrete per tanti, troppi cittadini che versano nelle stesse assurde condizioni. Oggi lo Stato intende farsi carico delle proprie responsabilità, rispondendo finalmente al grido di aiuto di quanti vivono le difficoltà economiche come un cappio al collo che stringe fino a portare alla disperazione e alla depressione, quando non addirittura, purtroppo, al compimento di gesti estremi. Con questo intervento di garanzia, lo Stato lancia un salvagente ai piccoli imprenditori per evitare che i creditori intacchino il loro patrimonio personale, consentendo di riuscire a salvare i propri beni oltre che la propria azienda; una misura, peraltro, premiante delle imprese sane e con prospettive di sviluppo in quanto la concessione della garanzia è condizionata alla sottoscrizione di un piano di rientro del debito tra banca e impresa beneficiaria che procedono a una rinegoziazione del precedente finanziamento, soprattutto relativamente alla sua durata. In questo modo, l'Italia entra di diritto nel novero dei Paesi più moderni in tema di sostegno alle imprese. imprese. Concludo il primo intervento che mi onoro di tenere in quest'Aula manifestando la mia assoluta convinzione e la mia più grande soddisfazione nel sostenere questo provvedimento che affronta con coraggio e determinazione i problemi che una pessima politica ha creato alla parte migliore e produttiva del nostro Paese. Per questo dico: mai più falliti per colpa dello Stato! *(Applausi

onorevole rappresentante del Governo, colleghi, la forza del nostro Paese è rappresentata dall'agroalimentare, dall'artigianato e dalle piccole e medie imprese. Compito ineludibile del Governo è migliorare il prestigio di tali peculiarità in modo da rendere l'Italia modello internazionale più di quanto non gli sia già riconosciuto. Agevolare la creatività, il gusto, la ricercatezza delle nostre produzioni è fondamentale per continuare sulla strada del primato. Il prestigio del nostro saper fare si accresce instaurando un continuo scambio di informazioni tra gli operatori dei settori e chi opera nelle istituzioni per stare al passo con i tempi, se non precorrerli, puntando all'innovazione combinata alla sostenibilità. La direttrice richiesta per dare sollievo ai diversi settori è la semplificazione delle normative e quindi, anche in agricoltura, è necessario porre attenzione e dare la giusta importanza a un settore primario per eccellenza e prestigio. L'agricoltura si sta rivelando un ramo della nostra economia di interesse crescente, soprattutto per i giovani con grado di istruzione alta, nonostante una serie di problematiche legate ai rischi di scarsa redditività, agli intralci burocratici e alla poca attenzione in sede europea, oltre all'ormai annoso dominio della distribuzione sulla produzione. Ma noi siamo qui, con il massimo impegno, per riequilibrare il settore, riconoscere agli agricoltori la giusta ricompensa per il lavoro svolto, mantenendo la consapevolezza sui pesanti e imprevedibili rischi a cui sono frequentemente soggetti, tra cui quelli climatici. Non è più trascurabile infatti la gestione del rischio delle avversità naturali in quanto queste si stanno estremizzando, procurando danni insostenibili per le aziende. Indispensabile è una più proficua ed efficace collaborazione fra Stato e Regioni nei rispettivi piani di sviluppo rurale, mantenendo ben delineate e tipiche le produzioni legate al territorio. Pur nella scia di una favorevole rinascita, ancora tanto lavoro ci aspetta, sia per quanto di nostra competenza sia in sede europea, in vista anche della programmazione PAC 2021-2027. È opportuno, quindi, un piano strategico nazionale in agricoltura da far pesare in sede comunitaria, che abbia come principale obiettivo una maggiore redditività per gli agricoltori, una maggiore coesione nel mondo agricolo e cooperazione fra piccole imprese. Nel decreto-legge semplificazioni poniamo i primi mattoni per andare incontro alle istanze degli operatori del settore agricolo. Di certo continueremo a confrontarci con tutti affinché non si smorzi la vitalità in atto, senza reprimere la qualità degli adempimenti a tutela di lavoratori e consumatori. Si vuole introdurre l'eliminazione di ripetitive compilazioni di documenti fra i vari uffici dando la possibilità di scambiarsi i dati; semplificazione nei rapporti di lavoro per tempi brevi, sia per accertamenti sanitari che per i pagamenti. Si vuol facilitare il riconoscimento della qualifica di agricoltore laddove vi siano una reale attività prestata e la passione per la coltivazione della terra. Da non trascurare é la premialità per aziende virtuose, in tema di retta applicazione delle norme e in termini di innovazione nell'accoppiata produttività e sostenibilità. favorire il rafforzamento degli strumenti di organizzazione delle OP per controbilanciare il potere dominante della distribuzione nella filiera agroalimentare; promuovere un più facile accesso al credito per le imprese agricole a minor interesse. In termini di trasparenza bisogna adoperarsi inderogabilmente sull'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine delle materie prime sulle etichette dei prodotti in vendita, in ogni sede; per una più rapida diffusione su larga scala di piattaforme digitali che vadano incontro alla semplificazione, unanimemente richiesta, e al minor consumo di carta, insieme all'installazione di reti di comunicazione ad alta velocità, oltre a una gestione più efficace che imponga un'accelerazione nel programma europeo dell'agenda digitale. Questi rappresentano solo alcuni punti che l'agricoltura nostrana dovrà affrontare nel futuro prossimo affinché diventi un comparto solido e competitivo. Nel panorama economico italiano è d'obbligo prestare attenzione all'agricoltura, settore basilare, anche se non rappresenta la voce più importante del prodotto interno lordo. Bisogna che si mettano in campo le migliori energie per far crescere un comparto primario che il mondo apprezza.

sulla quale voglio attirare l'attenzione dei superstiti di questa Assemblea che seguono la discussione generale. Soprattutto voglio attirare l'attenzione sia della maggioranza che dell'opposizione

e su questo attiro la vostra attenzione - c'è una vicenda relativa allo scorrimento delle graduatorie delle prove scritte del concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati al numero di 1.182), ossia la graduatoria dei cosiddetti civili. Qual è il contesto? Il Governo sta valutando di assumere 1.851 nuovi agenti di Polizia. Benissimo, non è questo il punto. C'è un «ma»: a sorpresa viene presentato un emendamento in base al quale verranno chiamati a svolgere le successive prove del concorso solo coloro che non abbiano compiuto i ventisei

del termine delle iscrizioni, e avevano conseguito la licenza media come titolo di studio. In forza dell'emendamento sul quale voglio attirare l'attenzione di tutti, migliaia di aspiranti poliziotti saranno - permettetemi il termine - buttati fuori dal concorso in virtù di una regola che viene creata e inserita successivamente al concorso. Gli aspiranti poliziotti in questione, che peraltro in questi giorni hanno cercato di denunciare anche attraverso le forme sindacali l'aberrante situazione, sono stati pregiudicati anche in passato - lo voglio dire - sempre a causa di di un criterio, non previsto neanche questo dal bando, e non vennero convocati a sostenere le prove fisiche perché l'amministrazione ne chiamò soltanto una piccola parte. Ma - come si dice - torniamo a bomba. Non si cambiano le regole del gioco in corso d'opera *(Applausi dal

del bando di 148 allievi di Polizia, chiuso - lo voglio ribadire - a maggio 2018, con un elenco di idonei non vincitori che puntavano a

in ballo, che puntavano allo scorrimento della graduatoria. Questo emendamento introduce nuovi criteri che di fatto eliminano buona parte

da altre persone che hanno ottenuto punteggi più bassi soltanto per una questione anagrafica. Mi chiedo e vi chiedo se un emendamento respinto in Commissione affari costituzionali, poi ripresentato, ritirato e modificato (ma in realtà non modificato affatto),

e reca, almeno nell'intento del testo originario e da quanto si evince dalla relazione introduttiva, disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, volte a superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato con la pubblica amministrazione. Si doveva dare un taglio alla burocrazia e facilitare la vita ai cittadini e alle imprese, ma nel lungo percorso al Senato il decreto, il decreto, di fatto, si è trasformato in un testo *omnibus*, arricchito di svariate norme, che vanno dalla riduzione dell'IRES per le *no profit,* ai 10 milioni per le famiglie delle vittime di Rigopiano; dagli NCC all'obbligo di distruzione degli ulivi affetti da Xylella, sino all'etichettatura. Ad allungare i tempi, c'è stato soprattutto il tema delle trivelle, che ha fatto procedere a singhiozzo i lavori delle Commissioni, sul quale poi è stato trovato un accordo che lascia un po' perplessi gli ambientalisti italiani. Ho presentato alcuni emendamenti che nelle Commissioni riunite purtroppo sono stati respinti. Avevo proposto una moratoria per le aziende agricole, anche nei precedenti provvedimenti, con una sospensione di ventiquattro mesi dei debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori in difficoltà. In caso di beneficio, gli stessi avrebbero potuto rateizzare i debiti Questa misura, sin dalla manovra di bilancio, è stata però dichiarata improponibile, nonostante l'articolo 1 del decreto-legge istituisca, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI. Un altro mio emendamento in materia ambientale, sempre respinto, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 41 del decreto Genova sui fanghi di depurazione. Le mie maggiori perplessità sulla novella approvata sono legate ai rapporti con la Carta costituzionale: in attesa di una revisione organica della normativa di settore - come aveva promesso anche il ministro Costa - occorre prestare attenzione affinché questa materia non impatti negativamente sul diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Il bene della vita e dell'ambiente meritano tutela e l'enorme aumento di limiti che abbiamo visto tenta di pregiudicare questi obiettivi. Del resto, anche l'Unione europea con le sue direttive ci invita alla prudenza e a una disciplina nell'utilizzo dei fanghi tesa a evitare effetti nocivi al suolo. Ho anche presentato alcuni ordini del giorno in materia di moratoria antiriciclaggio e trivellazione, anch'essi non considerati. La moratoria sulle trivellazioni, infatti, non precisa che saranno autorizzate 15 nuove rivelazioni, di cui 4 in mare e 11 su terraferma. La norma, infatti, salva dalla moratoria le istanze di concessione già in essere alla data di entrata in vigore della legge e anche le concessioni in scadenza verranno

dire che il senatore Pepe poteva fermare lo scempio in Basilicata, ma non l'ha fatto. Non ha impugnato la VIA che la Regione Basilicata aveva proposto attraverso una delibera, dimostrando così di essere più interessato al ristoro finanziario che alla tutela del nostro territorio. Ho accolto con favore, riguardo al comma 7, l'emendamento dei relatori sulla xylella, ma anche su questo tema ho presentato un emendamento sia in Commissione che in Aula. In questo decreto-legge si vogliono introdurre disposizioni per far fronte alla xylella e si vogliono deliberatamente autorizzare gli abbattimenti di alberi con una norma che addirittura introduce il carcere per chi si rifiuta di tagliare le piante; una violazione al diritto della proprietà privata e al nostro paesaggio che è tutelato dalla Costituzione. Lo stesso emendamento dei relatori ha previsto che questa norma di punibilità sia concepita in modo molto discrezionale. Giovedì faremo una conferenza stampa sul tema, perché lo stesso impianto normativo dovrebbe essere meglio implementato. Concludo dicendo che, in merito all'articolo relativo alla etichettatura, sarebbe stato opportuno, come chiedono i consumatori, inserire una norma che prevedesse anche l'indicazione dei residui tossicologici e non solo l'origine della materia prima. Mi riservo, su questo punto, di presentare una modifica nel primo provvedimento utile.

sta devastando alcune Regioni del Sud Italia, in principal modo la Regione Puglia. So che il ministro Centinaio sta lavorando e ha pronto un decreto, che molto probabilmente arriverà tardi, non certo per colpa del Ministro dell'agricoltura, ma per colpa di chi, negli anni passati, non ha voluto affrontare questa tematica. Oggi si è giunti alla stesura di un decreto che arriverà da quanto ci è dato sapere - a giorni e che affronterà (spero e sono convinto radicalmente) il tema dell'avanzata di questo flagello per l'olivicoltura del nostro Paese.

e nessuno è mai riuscito a risolvere il problema, oggi, molto probabilmente, riusciremo finalmente a dare una svolta verso la qualità, la trasparenza, la genuinità dei prodotti che arrivano sugli scaffali e sulle tavole dei nostri consumatori.

in questo Paese, diventasse, da pomodoro cinese, pomodoro prodotto in Italia. Quindi la massaia italiana, la signora Maria di turno,

Di questo dobbiamo essere orgogliosi, perché alla fine la qualità e la trasparenza si trasformeranno in una realtà anche reddituale, dando dignità alle risorse e al lavoro dei nostri bravi agricoltori.

ringrazio lei e per suo tramite ringrazio i colleghi che vorranno ascoltare questa considerazione in discussione generale, perché siamo ancora in tempo un'azione comune che impedisca un fatto gravissimo che rischia di consumarsi nei prossimi minuti. Mi riferisco al cambio in corsa

è troppo grave ciò che sta accadendo per giochicchiare alle responsabilità: nella scorsa legislatura, come lei ricorderà, Presidente, abbiamo approvato un provvedimento che riguarda i requisiti dei bandi che andremo a porre in essere da oggi in avanti, ma quello cui faccio riferimento è un bando aperto, è una graduatoria valida. Ebbene, sono così rispettoso di quest'Assemblea, anche quando sento cose lontane anni luce alla realtà, che vorrei unirmi all'appello del collega Paragone

è che avviciniamo all'idea della polizia e, dei servitori dello Stato indossando qualche divisa, in maniera secondo me discutibile, ma allontaniamo questa idea da quei ragazzi che avevano un solo intento, un solo sogno, una sola ambizione: quella di poter concorrere ad armi pari a diventare servitori dello Stato.

Presidente, colleghi, questa mattina mi sono svegliato in una Trento imbiancata e per noi trentini, che aspettavamo la neve, è certamente un motivo di soddisfazione. Quel bianco mi aveva anche portato a cercare di riflettere sull'intervento che avrei dovuto fare questa mattina, per essere il più possibile positivo, ottimista e costruttivo. Ho cercato quindi di coniugare la mia sensazione mattutina, determinata dal clima atmosferico che ho trovato nella mia città quando mi sono svegliato, mi sono svegliato, con i nostri lavori parlamentari. Nonostante la mia buona volontà e, come ho detto, la mia buona disposizione, ho fatto davvero fatica e anzi non sono purtroppo riuscito a trovare degli elementi che mi permettessero di parlare con positività

Pur criticando certi atteggiamenti anche di parte dell'opposizione, che non aveva avuto rispetto delle istituzioni,

cioè di essere il più possibile coerenti con un programma di serietà, nel quale le istituzioni siano davvero rappresentate in modo corretto. La correttezza sta certamente nel rispettare il voto nelle Commissioni, nell'intervenire senza offendere nessuno, nel non fare gesti plateali, come sono stati fatti anche in quest'Aula, ma la correttezza sta anche, da parte di chi ha l'onere e l'onore di amministrare il Paese,

delle semplificazioni nella sua vita, nel suo agire nell'impresa e nella propria attività professionale. Ebbene, questo si aspettano i nostri elettori, gli elettori della destra che rappresentiamo, ma anche gli elettori della sinistra e del centro, di chi sta sopra e di chi sta sotto;

lontane dalla realtà, che è preoccupata dall'approssimarsi delle elezioni europee e quindi è preoccupata di non essere pienamente coerente con le

esasperato, perché per bloccare la crescita e lo sviluppo, nell'ottica della decrescita felice, ovviamente bisogna andare verso l'ambientalismo esasperato, che è ben altro rispetto all'ambientalismo e alla tutela dell'ambiente.

da parte di tutti, di andare in una direzione più coerente, non tanto con le promesse, quanto con quella serietà, quella coerenza e quelle regole che devono improntare i nostri lavori parlamentari.

onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, probabilmente non impegnerò tutti e dieci i minuti e non lo farò per una questione di economia procedurale, perché stiamo attendendo l'esito del giudizio di ammissibilità sugli emendamenti e probabilmente rischieremmo di discutere di questioni e di argomenti che, di qui a qualche minuto, saranno dichiarati inammissibili per estraneità di materia. Cercherò, quindi, di contenere il mio intervento sui punti di questo decreto-legge, tralasciando gran parte delle innovazioni che sono state introdotte, a mio modesto avviso anche inopportunamente, in corso di causa.

una rigida attinenza ai temi del decreto-legge e poi presentare un numero così elevato di emendamenti. Il senatore Pepe, che pure ha seguito, come noi, i lavori di Commissione, deve darci atto - su questo chiamo anche, se possibile, a testimoniare i due Presidenti delle Commissioni - che proprio su espressa richiesta del Gruppo Forza Italia, nella persona del senatore Mallegni, è stato richiesto ai Presidenti di fare una valutazione rigida e non flessibile sui principi della ammissibilità degli emendamenti, a partire da quelli di Forza Italia. Abbiamo chiesto ai Presidenti di fare un lavoro stringente, coerente a quello che era il testo iniziale del decreto-legge, anche se fossero caduti emendamenti presentati da Forza Italia. Questo sta a dimostrare che noi le idee le avevamo chiarissime. E ci dispiace prendere atto che, nonostante il Presidente del'8a Commissione, subito dopo le audizioni, abbia dichiarato che si sarebbe opposto a che questo provvedimento diventasse un *omnibus*, un *omnibus*, si è verificato esattamente il contrario: questo decreto-legge è diventato un *omnibus* ed è diventato un espediente per aggirare i presupposti di legge per ottenere la decretazione d'urgenza. Si chiede la decretazione d'urgenza per argomenti improcrastinabili improcrastinabili e poi, durante la legge di conversione, vi si inserisce di tutto e di più, scavalcando anche le legittime prerogative dei parlamentari, che hanno diritto a discutere e ad approfondire nei tempi regolamentari le varie proposte di legge. Questo per amore di verità. Dobbiamo dare atto, pur nel complessivo giudizio negativo su questo decreto-legge, di qualche raggio di sole: poca roba, ma piuttosto che niente, meglio piuttosto, come diceva un mio maestro di vita e di professione. Abbiamo accolto immediatamente la richiesta del Governo e della maggioranza di espungere dagli emendamenti tutti quelli che riguardavano la materia degli appalti, perché è giusto che sul tema ci sia un intervento organico e strutturale, con i tempi e con i modi dei Regolamenti parlamentari, che possano innovare e rinnovare il settore. Dobbiamo dire anche che, grazie al nostro intervento, sono stati ritirati emendamenti che riguardavano le modifiche al codice di procedura penale. qualche giorno fa c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario e il Ministro della giustizia ha riproposto il suo programma, dicendo che entro il 31 dicembre 2019 sarà in grado di presentare la riforma - beato lui - del codice di procedura penale e anche quella del codice di procedura civile. Se questo è vero, non si capiva per quale motivo in questo decreto-legge, peraltro con un'estraneità assoluta di materia, si dovessero inserire elementi di modifica al codice di procedura penale. prendiamo atto con favore: la maggioranza, *melius re perpensa*, ha ritirato tutti questi emendamenti. Siamo stati soddisfatti

un altro aspetto positivo, che evidenzia la disparità di trattamento che a volte viene messa in atto dai rappresentanti della maggioranza. Avevamo presentato un emendamento, a mia prima firma, con il quale chiedevamo d'inserire nell'accesso al fondo di solidarietà anche i professionisti in difficoltà e non soltanto le aziende. Anch'essi, infatti, a seguito del ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, si trovano in gravi difficoltà. Detto emendamento è stato respinto,

alla norma, se non aiutiamo il settore dell'olivicoltura pugliese stabilendo un fondo straordinario di sostegno ai nostri olivicoltori e nominando un commissario straordinario che possa sovrintendere a tale iniziativa. FI-BP).* E dove prendiamo i soldi? Dal reddito di cittadinanza, che non partirà mai in questo Paese: almeno serviranno a garantire un settore importante del Mezzogiorno d'Italia e della Puglia. Non siamo assolutamente soddisfatti di come avete affrontato il tema delle trivelle, prendendovi in giro da soli perché non è vero che avete stabilito una moratoria:

per sanare le difficoltà all'interno di questa maggioranza. Avete utilizzato lo strumento del decreto-legge per una ritorsione politica nei confronti dei rappresentanti dell'opposizione, andando a toccare il consiglio di amministrazione dell'ENAV con un provvedimento

Ultima, ma non per ultima, è la vergogna che è stata già citata dalla collega Rauti e dal collega Richetti: non è possibile cambiare le regole in corso d'opera, deludendo i cittadini che hanno svolto un concorso e che, anche se non l'hanno superato, sono stati dichiarati idonei e, in quanto tali, sono

faccia grazia, per dire che questo provvedimento, purtroppo, seguirà la sorte di tutti gli altri. Il decreto dignità dovuto procurare lavoro: è vero che c'è stato un aumento delle occupazioni a tempo indeterminato, è però aumentata la disoccupazione, perché gli imprenditori sono stati disincentivati dall'assumere a tempo determinato. La legge di stabilità ha dimenticato il Mezzogiorno: meno investimenti, meno credito d'imposta, meno superammortamento, meno ammortamento e lo spazzacorrotti non è altro che un provvedimento a favore dei corrotti. Non devo citare quello che vi è stato detto all'inaugurazione dell'anno giudiziario, dove non c'è stata una parola a favore di questo provvedimento. Mai, come in questo caso, tutto il mondo giudiziario, giurisprudenziale, dei professionisti del diritto e degli avvocati è stato unanime nel dire che questa è ed è stata una porcheria! E non basta la norma per snellire le procedure per le carceri, perché servono i denari. Di qui a qualche anno, con tutte le eccezioni che avete creato e con tutta l'inaccessibilità che avete creato nei confronti delle forme alternative alla detenzione, avremo 30.000-40.000 detenuti in più, che non sapremo dove collocare e credo che voi non abbiate idea di come si faccia ad affrontare questo problema. Comunque, noi siamo qui, in attesa che il popolo italiano - sovrano, come sempre - si decida e possa finalmente dare un giudizio definitivo su questo Governo e su questa maggioranza. Buona fortuna.

intervengo con rinnovato orgoglio per le decisioni prese dal Governo e dalla maggioranza. Ancora un provvedimento importante, ancora un'azione incisiva per le fasce deboli, rivolgo al senatore Vitali - le imprese, l'ambiente, l'energia e anche l'istruzione. Le Commissioni hanno dato un prezioso contributo; ringrazio i senatori e i collaboratori legislativi, senza dimenticare i funzionari, che in maniera pregevole hanno concorso al miglioramento del testo in esame, che semplifica i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Faccio solo qualche sottolineatura sulla rilevante fase emendativa. Assicurare sostegno alle aziende in credito con la pubblica amministrazione che faticano a restituire le rate è certamente una misura giusta, equa e di buon senso, così come permettere di continuare ad abitare gli immobili pignorati. Bene il rinnovo della restituzione del prestito ponte: parliamo di Alitalia; poi un giorno le opposizioni ci spiegheranno il senso di quella bellissima e indovinata battuta «allacciate le cinture», indimenticabile direi. *(Applausi agroalimentare finalmente arriva l'etichetta con l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza. Bene anche la norma che facilita i professionisti non organizzati in collegi o ordini. Bene il far fronte alla contingente carenza di medici, così come l'assunzione di dirigenti scolastici, una misura necessaria, che anticipa importanti provvedimenti nel mondo dell'istruzione. Vorrei però soffermarmi più dettagliatamente su due aspetti: il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (le trivellazioni, per capirci) e le misure di sostegno ai familiari delle 29 vittime di Rigopiano. Entrambe queste misure sono frutto di battaglie del MoVimento, anche private, portate avanti personalmente con il sostegno e la condivisione di tutti i colleghi del MoVimento e anche della maggioranza. Ho bene in mente l'incontro con un gruppo di persone che ha visto la propria vita stravolta dal tragico evento di Rigopiano, Farindola, Abruzzo. Ricordo la loro emozione e ricordo il peso delle loro parole, che, come rappresentante delle istituzioni, ho sentito molto forte sulle mie spalle: «senatore, siamo stati abbandonati». Rigopiano è un dolore ancora aperto, se è vero, come è vero, che c'è un'inchiesta *bis* a carico del prefetto e di altri sei esponenti della prefettura per depistaggio e frode processuale. Già nella legge di bilancio, così come nel decreto fiscale, avevamo provato a inserire misure a sostegno di quelle famiglie. Oggi finalmente ci riusciamo, grazie alla sensibilità e alla concretezza del Governo del cambiamento, che ha inteso intervenire con uno stanziamento di 10 milioni di euro. Oggi sento di poter dare una risposta a quelle persone che ho incontrato: non siete soli, siamo al vostro fianco, abbiamo svolto il nostro dovere. Vengo alle trivelle. Nei giorni scorsi siamo stati accusati di molte cose; per alcuni saremmo quasi diventati «Sì Triv»: una follia. Lo ribadisco a gran voce, senatore Vitali, mi ascolti: noi siamo e resteremo contro le trivelle. Chi vi parla è il primo firmatario di un disegno di legge recante norme per il divieto dell'utilizzo dell'*air gun*: presto battaglieremo affinché il ricorso all'*air gun* diventi una pratica illegale. Anche le pietre sanno che governiamo avendo sottoscritto un contratto con la Lega: questo significa, tra le altre cose, che occorrono mediazione politica e compromesso parlamentare. L'emendamento approvato prevede l'adozione del Piano delle aree: ci diamo un tempo congruo (18 mesi), accompagnato da una speciale moratoria fino all'approvazione del Piano stesso, moratoria che si sostanzia nella sospensione dei procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi e la messa in regime di sospensione temporale per i permessi di prospezione e ricerca in essere,

abbiamo aumentato - e era ora - i canoni annuali di ben 25 volte: il solo gettito, a situazione attuale, passerebbe da circa 1.330.000 euro a ben 33 milioni di euro. Si potrebbero generare delle richieste di risarcimento? Certamente, ma siamo pronti anche a questo: abbiamo già risorse sufficienti e comunque la possibilità di rimodulare quindi una certezza ai cittadini: sicuramente non pagheranno loro. L'emendamento blocca 38 permessi vigenti e 85 istanze pendenti.

Concludo manifestando ancora una volta la soddisfazione per le misure contenute in questo decreto-legge e anche perché stiamo procedendo a testa alta. La maggioranza tutta sta lavorando incessantemente e con decisione su un percorso immaginato da tempo che va nella direzione sottoscritta nel contratto. Qualche mese fa tutto questo sembrava impossibile; invece stiamo brillantemente cambiando la storia del Paese. Giorni or sono, e concludo Presidente, affermai proprio in quest'Aula che stavamo andando alla grande. Oggi lo confermo ed esorto tutti i colleghi di maggioranza ad andare avanti con risolutezza e con determinazione verso l'ormai inevitabile e agognato cambiamento.

*dal Presidente del Consiglio dei ministri* *e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali* «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».

le piccole e medie imprese che hanno debiti consolidati verso lo Stato. Si introducono norme per cui chi

sul volo, la nostra non li fa. Vuol dire che è stata gestita male. Se vogliamo stare accanto alla compagnia di bandiera, e sappiamo che

regolazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali (DURC), abbiamo allungato i tempi.

intraprendere la propria attività in una ZLS, incontra una serie di contrasti burocratici e amministrativi veramente complessi. Andiamo loro incontro.

etichette facilmente leggibili, che permettono di tracciare i prodotti e sapere se ciò che mangiamo è prodotto in Cina, in Uzbekistan o chissà dove e che può essere composto da organismi geneticamente modificati.

nel momento in cui arriva il pignoramento sono costrette a lasciare la casa, anche se per due o tre anni non viene venduta. Introduciamo quindi delle regole affinché queste persone

carcerario. Sappiamo che le carceri sono sovraffollate, abbiamo avanzato delle proposte per

abbiamo fatto delle scelte, certamente molti NCC non ne saranno contenti, ma sappiamo che c'erano delle irregolarità per alcune Province e per alcune Città metropolitane e Roma è una di queste. Sicuramente a livello nazionale con queste regole non andremo incontro a tutte le esigenze specifiche, ma

trivelle credo che larga parte di questo Parlamento sia d'accordo. Abbiamo fatto un'opera d'arte accettando le esigenze del MoVimento 5 Stelle, delle forze ambientaliste di questo Paese, che erano stanche di vedere puntare tutto sul fossile e,

il programma energetico. Innanzitutto lo ridefiniamo e ci diamo del tempo per verificare. Colleghi, non so se avete visto cosa è successo con le auto

FI-BP)*. Uno degli emendamenti riguarda le derivazioni idroelettriche, che vengono normate, nel caso in cui, a seguito di vetustà, esse non siano più utilizzate e quindi vengono messe in capo alle Regioni: mi sembra una previsione giustissima. Siamo intervenuti sull'ineleggibilità degli avvocati, che era una questione sospesa da tempo. Abbiamo poi introdotto una serie di semplificazioni importanti, dal punto di vista contabile. Se volete, faccio tutta la lista delle semplificazioni...

Infine siamo intervenuti sulle questioni della disabilità, che credo siano importantissime per le persone disabili che vivono nel Paese.

che questo procedimento e questa lunga avventura, che abbiamo affrontato tutti insieme nelle Commissioni riunite, costituiscano un esempio lampante delle difficoltà che possono avere i cittadini

si può salvare e cosa invece non si può salvare. Ci sono tantissime disposizioni all'interno di questo decreto che sono buone e che erano, fra l'altro, condivise dalla maggioranza e anche dalle opposizioni che ovviamente non abbiamo potuto portare a termine. Ce ne sono tante altre, ritenute anche urgenti - e quindi ritorniamo al senso del decreto d'urgenza - che siamo riusciti ad inserire. Altre però, ritenute urgenti dalla dalla quasi totalità dei commissari, probabilmente non arriveranno alla fine della storia di questo decreto-legge. Questa è la differenza che forse i cittadini non riescono a cogliere. Giustamente, dopo tanti anni in cui si attendono delle soluzioni, le si vorrebbero subito, nel primo provvedimento utile. Per fortuna noi, come mi auguro, avremo davanti del tempo per procedere con altre semplificazioni e altri provvedimenti assolutamente necessari per questo Paese. Noi ci abbiamo provato. Quando questa mattina ho detto che siamo stati accusati di aver lavorato troppo, l'ho detto in modo ironico ma il concetto era reale, nel senso che abbiamo cercato noi, ma anche le opposizioni, di inserire tanti argomenti e di risolvere in una volta sola tantissimi problemi che la gente si aspetta siano risolti il prima possibile. Mai mi sarei aspettata di fare un lavoro simile,

su alcune tematiche politicamente molto rilevanti, di essere costretti gli uni con gli altri a tapparci il naso per votare i rispettivi emendamenti e, come ho detto in quella sede e ripeto anche qui, mai nessuno qui si è tappato il naso e mai lo farà, perché noi lavoriamo insieme e discutiamo fino a quando non arriviamo ad un risultato condiviso.

che tutto il lavoro fatto nelle Commissioni riunite con la maggioranza, ma anche con le opposizioni, non verrà perso, anche ciò che non arriverà alla fine dell'esame del provvedimento. Ci saranno molte altre tematiche su cui confrontarci. Comunque abbiamo sviscerato talmente tante ci siamo anche conosciuti meglio, anche, perché abbiamo lavorato con i membri di altre Commissioni e abbiamo capito quali sono le sensibilità di ognuno e siamo arrivati ad un risultato. Non posso, quindi, che essere orgogliosa del gruppo che si è creato

intervengo dopo aver sentito per alcune ore, da questa mattina, gli interventi dei senatori di maggioranza e di opposizione, per ribadire alcuni dei passaggi significativi del provvedimento in discussione. Anch'io in questi giorni sarebbe più corretto dire in queste settimane - ho partecipato in maniera praticamente costante ai lavori delle Commissioni riunite e devo dire che mi trovo assolutamente d'accordo con quanto detto dai relatori dai relatori e anche dal relatore di minoranza, riguardo il lavoro fatto in queste lunghe, a volte lunghissime giornate. Il provvedimento in discussione sicuramente non era semplicissimo, come tutti i provvedimenti che derivano da decreti che normalmente, appunto, rispondono a delle urgenze e che poi, nel e che poi, nel passare dei mesi, nel corso della loro applicazione definitiva, devono affrontare inevitabilmente situazioni nuove che si sono venute a creare e quindi con la necessità magari di rivedere, migliorandole, alcune delle cose che erano state previste ed eventualmente

marginale nell'entità, ma non marginalissimo: c'è anche una sorta di tassa annuale da pagare solo per il fatto che questo sistema esiste. Il Sistri era nato forse in un momento in cui si aveva un'esagerata

affidarsi a cose fantasiose, terze e spesso improbabili per risolvere ogni problema; basterebbe applicare con più serietà e partecipazione, da parte di tutti gli attori della società, un corretto comportamento in tutti i passaggi di tipo aziendale.

tranquillamente sotto controllo anche senza il Sistri. Io credo che le cose gravissime che sono accadute, e che probabilmente accadono ancora nel Paese per quanto riguarda la gestione non corretta dei rifiuti non siano da imputare a marginalità che con un sistema digitale potremmo andare a controllare; credo semplicemente che ci siano dei passaggi macroscopici che in tanti fanno finta di non vedere, altrimenti alcune cose che accadono non dovrebbero assolutamente verificarsi. Per quanto riguarda il discorso relativo agli appalti pubblici, anche qui è stata sottolineata l'importanza di andare verso una revisione che porti a una semplificazione di tutto il codice degli appalti; non certo perché si vogliano o si voglia rendere il sistema più permeabile ad attività illegali, ma perché non si deve, come spesso si fa, andare da un eccesso al suo opposto. Non si può pensare di ingabbiare qualunque tipo di lavoro pubblico, anche di piccola entità, con regole che non solo sono estremamente complicate da applicare e allungano moltissimo i tempi necessari per svolgere le opere pubbliche, ma che spesso negli ultimi tre anni hanno talmente spaventato i funzionari pubblici che, nel dubbio, nella maggior parte dei casi, si preferisce aspettare e non fare nulla per essere sicurissimi di qualunque passaggio. Il risultato è che per fare un semplice marciapiede o 50 metri di fognatura ci vuole non più qualche mese (come era ovvio e logico fino a qualche anno fa) ma addirittura qualche anno. In un momento in cui il Paese ha bisogno di un po' di economia reale credo che i lavori pubblici già finanziati, con risorse economiche disponibili, debbano essere fatti nella maniera più veloce e altrettanto regolare possibile; credo che questo sia uno degli obiettivi che tutti insieme dobbiamo raggiungere. In questo senso questa maggioranza e questo Governo, nella manovra finanziaria appena terminata, comunque sbloccato una quantità di risorse che, pur se in assoluto non sono epocali, comunque sono assolutamente importanti. Esse hanno già prodotto, negli ultimi mesi dell'anno appena passato

delle nostre aziende che lavorano anche negli appalti e nei lavori pubblici), dando effettivamente un contributo significativo, ma soprattutto immediato, al mantenimento del PIL del Paese, che sappiamo essere uno dei problemi che tutti insieme dobbiamo dobbiamo affrontare. Quindi quel po' di semplificazioni che sono state messe in campo sono assolutamente fondamentali per poter velocemente dar luogo ai lavori pubblici che abbiamo in mente di sbloccare. Nel ricollegarmi ad alcuni interventi che sono stati svolti, devo dire che io mi sento di appartenere a un Paese normale, dove la normalità è quella di persone che fanno bene, onestamente e correttamente il proprio lavoro (se lavorano in aziende) la propria attività pubblica (se sono transitoriamente amministratori locali). Quindi non è corretto tarare qualunque intervento solo sulla parte marginale di chi è fuori dalle regole, mettendo in difficoltà la stragrande maggioranza di chi invece vive tranquillamente, non perché la legge glielo impone, ma perché è così come persona (insieme appunto alla maggior parte delle persone) e svolge con tranquillità, serenità e onestà intellettuale il proprio mestiere. ognuno può pensare degli altri quello che pensa di sé; ma credo che la maggior parte di noi qui presenti sia convinta che l'Italia sia fatta da persone serie, oneste e corrette. Per quanto riguarda il discorso delle aziende in crisi, credo che anche da questo punto di vista siano stati svolti degli interventi importanti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a due fenomeni altrettanto gravi. che devo dire più che grave è veramente incredibile - è quello delle aziende che hanno corso il rischio di fallire nella propria attività, o addirittura sono state obbligate a chiudere, non per incapacità amministrativa propria o per mancanza di lavoro e di capacità di far rendere il proprio lavoro, ma semplicemente perché creditrici nei confronti dello Stato. In particolare, di fronte ad uno Stato che, da una parte, richiede con

traversata, dandole il colpo di grazia e facendola chiudere, dobbiamo invece tendere il braccio, cercando di farle completare la traversata e farla ripartire a nuova vita. Ci sono poi gli ultimi due argomenti importanti

illustrato da chi mi ha preceduto. Voglio solo aggiungere qualche considerazione: la maggior parte delle centrali idroelettriche, quindi quelle veramente a impatto zero per definizione,

la questione trivelle, credo sia chiaro a tutti che il movimento politico cui mi onoro di appartenere ha delle idee sulle questioni economiche abbastanza precise che non ha mai nascosto ed ha sempre portato avanti. Questo non significa che sull'altare dell'economia, dei soldi e dello sviluppo momentaneo si debba sacrificare qualunque altra cosa. Il Paese bellissimo in cui tutti noi abitiamo, infatti, è un Paese cui ovviamente vogliamo particolarmente bene

alle concessioni. Non credo banalmente - e dico due numeri che dovrebbero da soli far riflettere - che un Paese possa dare in concessione più o meno 30.000 chilometri quadrati, cioè una volta e mezzo la Lombardia, e portarsi a casa meno di due milioni di euro. Credo che ci sia qualcosa che non va e che ogni altro discorso semplicemente si commenti da solo. Chiedo solo un minuto per entrare nel merito politico di una questione che, ovviamente (ma è giusto perché ognuno fa il proprio mestiere) ha riempito i giornali e fatto i titoli nelle scorse settimane:

ad una conclusione, non si arriva ad un compromesso ma, dopo un'adeguata riflessione, ad una soluzione equilibrata che normalmente tiene conto delle esigenze di tutti e probabilmente tiene conto della media del pensiero del Paese.

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha attentamente valutato gli emendamenti, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo

Il decreto-legge in esame si compone di 12 articoli (norme in materia di imprese, restituzione del finanziamento Alitalia, modifiche al codice degli appalti, edilizia penitenziaria, informatizzazione, istruzione e ricerca, trattamento economico del personale della pubblica amministrazione). Ha pertanto un contenuto plurimo, secondo la definizione ricorrente nella giurisprudenza della Corte per provvedimenti analoghi. Risponde quindi alla finalità di introdurre, come specificato nel titolo e nelle premesse, «disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», al fine di superare

la Presidenza, come indicato dalla giurisprudenza dalla Corte costituzionale (recentemente, ad esempio, nella sentenza n. 32 del 2014) ha esaminato la proponibilità degli emendamenti valutandone il collegamento con la «*ratio* dominante» del decreto-legge. Sono stati pertanto ritenuti proponibili gli emendamenti che introducono misure di sostegno, semplificazione, modernizzazione per i soggetti economici, per la pubblica amministrazione in generale nonché per l'azione pubblica, così come le proposte emendative concernenti modalità di semplificazione per l'esercizio o la tutela di posizioni giuridiche soggettive, in quanto in essi si ravvisa la necessaria coerenza rispetto al contenuto e alle finalità del provvedimento d'urgenza. Risultano in primo luogo improponibili gli emendamenti che prevedono il conferimento di deleghe legislative. Sono state inoltre ritenute estranee all'oggetto del decreto-legge le proposte di modifica recanti disposizioni che non si traducono in misure di semplificazione o sostegno, ovvero che non siano riconducibili ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge

1.34, 1.44, 1.0.500, 2.1000, 3.47, 3.500, 3.0.81, 3.0.136, 3.0.700, 4.3, 4.0.1000, 8.500, 8.0.3, 8.0.500, 9.0.41, 9.0.500, 10.0.1000, 11.0.43, 11.0.95, 11.0.172, 11.0.500, 11.0.600, 11.0.1000. Gli altri emendamenti approvati dalle Commissioni riunite risultano invece improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in conformità ai criteri sopra enunciati. Risultano inoltre improponibili i subemendamenti ai predetti emendamenti approvati dalle Commissioni riunite: 3.500/700 11.0.43/408 e 11.0.43/409; 11.0.1000/500. Relativamente ai subemendamenti all'emendamento 11.0.500 risultano proponibili i soli emendamenti 11.0.500/8 e 11.0.500/9; gli altri subemendamenti a tale emendamento sono tutti improponibili.

Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per esprimere - a seguito di queste sue determinazioni - una richiesta, ovvero che i lavori per l'esame degli emendamenti riprendano domattina, in maniera tale che sia consentito a tutti i Gruppi di poter prendere in esame nel dettaglio le sue determinazioni e avere a disposizione un fascicolo completo e ordinato, come già più volte richiesto. In realtà, dico questo premettendo un apprezzamento da parte del Gruppo Partito Democratico rispetto alla sensibilità che lei ha mostrato

alla confezione di un almanacco di forzature e incostituzionalità - alle quali oggi si è aggiunta anche la pratica dell'auto-ostruzionismo della maggioranza - che rendono anche questa una pagina non bella per i nostri lavori. abbiamo più volte sottolineato quanto questo provvedimento si stesse allontanando dalle caratteristiche e dai requisiti che deve avere un decreto-legge. Come già più volte ricordato dalla Corte costituzionale nel nel 2007 e nel 2008, il tema dell'omogeneità è determinante per stabilire se un decreto-legge è costituzionale o no, perché è legata alla sua omogeneità la motivazione per cui il decreto stesso viene formulato dal Governo, ovvero la presenza di condizioni straordinarie ed urgenti.

Dobbiamo dire grazie anche al fatto che finalmente si arriva ad affrontare, con la sua determinazione, signor Presidente, un tema che avevamo segnalato attraverso il presidente Marcucci in più di un'occasione durante la Conferenza dei Capigruppo. Non è possibile

aperte", della vita dei cittadini, delle imprese, di comparti interi cui si riferiscono aziende quotate in borsa, il tutto addirittura in attesa che a un certo punto il Presidente, in maniera saggia,

quando avremo coscienza complessiva dei lavori che dovremo affrontare nell'esaminare gli emendamenti e anche in ragione di un'esigenza del Partito Democratico di poter svolgere, nel corso di questo pomeriggio, una riunione del Gruppo che ci consenta di riesaminare un provvedimento diverso da quello che è stato incardinato questa mattina

anche noi chiediamo di poter avere un tempo congruo per poter riesaminare il tutto. Certamente apprezziamo il lavoro che lei ha fatto, ma credo anche che abbiamo la necessità di una serie di riflessioni, anche per il futuro.

anche da oggi, si inauguri finalmente una prassi nuova, molto allineata ai pronunciamenti della Corte costituzionale, allo spirito costituzionale e quindi, soprattutto in materia di decreti-legge, di tornare ad avere una possibilità vera almeno di omogeneità. È chiaro che

perché lei sa, Presidente, che i Presidenti di Commissione rivendicano sempre la loro autonomia - e questo lo prevede anche il Regolamento - per quanto riguarda le dichiarazioni di ammissibilità, ma poi ci troviamo in questa situazione. Alla fine siamo stati

la ragione, tra l'altro, del sovradimensionamento degli emendamenti. È evidente che, nel momento in cui maggioranza e relatori presentano emendamenti, l'opposizione presenta i

deve portare a casa. Questo modo di procedere ci sta portando a perdere non solo tanto tempo, Presidente, ma anche credibilità nel lavoro di tutto il Parlamento.

la discussione sul provvedimento nei canali delle regole stabilite, anche dalle norme importanti e dalle decisioni della Corte costituzionale che lei ci ha letto prima di riferirci l'elenco degli emendamenti ammissibili.

Tutti i nostri componenti delle Commissioni hanno sottolineato questo aspetto in modo costante, rilevando l'estraneità per materia di molti emendamenti

in gran parte inutile, che avrebbero potuto essere organizzate molto meglio: si sarebbero potuti, probabilmente, evitare i ritardi della settimana scorsa e una serie di cose che rendono più difficile - dunque meno efficace - il lavoro del Senato. Alla luce di tutto ciò e del fatto che lei ha annunciato che le ammissibilità o le inammissibilità per quanto riguarda gli altri emendamenti, a parte quelli approvati dalle Commissioni riunite, saranno rese note nelle prossime ore,

numerosi altri (immaginiamo): è evidente che i criteri che lei ha citato, applicati all'insieme degli emendamenti, daranno luogo a molte dichiarazioni di inammissibilità.

ed è necessario accettare, qualsiasi essa sia, la pronuncia della Presidenza rispetto alle improponibilità e alle inammissibilità. Esistono Esistono senatori che presentano emendamenti che vengono dichiarati inammissibili, così come esistono partiti politici che presentano ricorsi alla Corte costituzionale che vengono dichiarati inammissibili, esattamente come successo per il ricorso del Partito Democratico,

di analizzare le inammissibilità. Noi proponiamo, però, di sospendere la seduta per dare tempo alla Presidenza di comunicare le successive inammissibilità, anche fino alle ore

di procedere con delle semplificazioni. Condividiamo la proposta del collega Patuanelli perché evidentemente abbiamo bisogno anche noi del tempo necessario per valutare tutti gli emendamenti. In attesa anche di capire quali emendamenti, tra quelli presentati e non approvati nelle Commissioni

Naturalmente, oltre a ringraziare lei, ringrazio anche tutti i commissari di opposizione che per venti giorni hanno mantenuto le loro posizioni nelle Commissioni riunite e in Commissione bilancio e hanno reso possibile

venga discusso compiutamente. Noi conosciamo solo in parte ciò che è rimasto dalla lettura che lei ci ha dato delle improponibilità,

tempo su questo provvedimento - che comunque abbiamo già concordato - nella giornata di oggi e di domani. Quindi non limitandoci, così come è stato proposto dalla maggioranza, alle dichiarazioni di voto e al voto finale nella giornata di domani, bensì alla discussione di ciò che è rimasto di questo provvedimento rispetto al lavoro fatto finora. Se non c'è nessun altro che desidera intervenire, direi qual è il mio pensiero. Ritengo di sospendere la seduta fino alle ore 18, in modo che possiate verificare gli emendamenti che sono stati ammessi

alle ore 18,21)*. Onorevoli colleghi, l'ulteriore elenco degli emendamenti non approvati dalle Commissioni riunite 1a e 8a e dichiarati improponibili è in distribuzione.

Signor Presidente, anche noi accogliamo l'invito del collega Patuanelli per rinviare a domani l'analisi degli emendamenti. Anche noi utilizzeremo il nostro tempo residuo per l'illustrazione di quelli che saranno sopravvissuti alla tagliola

Chiedo quindi a lei e agli Uffici di verificare le motivazioni di una tale inammissibilità, trattandosi di emendamento perfettamente coerente con il testo da emendare: entrambi si riferiscono a modifiche della legge n. 113 del 2017, intervengono su due articoli diversi,

emendamenti da loro prospettati come oggetto di ripensamento devo dire che ho a lungo riflettuto su tutti, uno per uno, in maniera molto meticolosa e,

nuova finestra"). L'informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Venezuela avrà luogo mercoledì 30 gennaio alle ore 18.

Presidente, colleghi senatori, mi pregio di comunicare la situazione di grave emergenza in cui versano le aziende sanitarie della Regione Toscana

Sono giunte certamente anche a voi le notizie in merito all'ultima controversa vicenda delle indagini della procura e della Guardia di finanza di Firenze su concorsi truccati per favoritismi personali nelle assunzioni di medici nei ruoli di primari di alcuni reparti del policlinico fiorentino di Careggi; la notizia di un altro scandalo giudiziario che ha coinvolto l'ospedale di Prato, per il quale l'indagine della procura pratese si è concentrata su una pratica consolidata di esenzione abusiva di *ticket* su cui invece il *ticket* era previsto, e sull'esercizio di attività ambulatoriali clandestine. Altre inchieste giudiziarie vedono o hanno visto protagonisti i vertici delle direzioni ASL toscane (Massa, Siena e la nuova macro-ASL Toscana Nord-Ovest), con accuse che spaziano dalla corruzione agli ammanchi di bilancio, fino ai concorsi truccati. Episodi più o meno Episodi più o meno eclatanti di malfunzionamenti della macchina amministrativa e burocratica, nonché carenze nell'erogazione di servizi e dispositivi sanitari per malati gravi, oltre all'ormai cronica insufficienza di personale medico-sanitario e ai problemi strutturali riscontrabili in molti ospedali, anche di recentissima realizzazione, sono prassi in tutta la Toscana. Preso atto di quanto detto, chiedo di adoperarsi affinché in tempi ragionevoli si proceda verso una sistematica attività ispettiva nelle ASL della Regione Toscana e, ove si ritenga necessario e opportuno,

mi spiace molto prendere la parola sempre a fine giornata per ricordare quelle che io considero oggettivamente delle gravi inadempienze da parte del Governo,

trattano problemi molto concreti che riguardano: bambini che sono stati - a mio avviso - ingiustamente allontanati dalla famiglia; alcuni aspetti profondamente problematici nella gestione della Croce Rossa; Croce Rossa; le dinamiche concrete della scuola e anche in ordine a una serie di figure professionali; la sanità, la gestione di farmaci e, in particolare, di farmaci orfani che risultano introvabili sul territorio.

più concrete del dialogo dei cittadini con l'attività politica e con le istituzioni. A me sembra sinceramente che questo Governo del cambiamento, perlomeno in merito alle risposte alle interrogazioni, sia di gran lunga peggiore dei Governi delle legislature precedenti. Non è mai capitato di avere una sequenza talmente lunga di domande e di interrogazioni concrete, documentate e poste da interlocutori che si aspettano una risposta. Penso a tutti quelli delle malattie rare - c'è stato sabato scorso il convegno sull'eosinofilia

perché richiami il Governo - che non si sa esattamente perché debba avere tanto da fare e più da fare di Governi precedenti, considerati anche i vuoti a cui assistiamo nella gestione del lavoro ordinario delle Commissioni

colleghi, prendo la parola su una vicenda che, qualora venisse confermata, si configurerebbe come episodio di assoluta serietà e da condannare senza se e senza ma. notizie di stampa, secondo le quali, nel corso di un incontro di calcio nella categoria di promozione, il direttore di gara avrebbe insultato un portiere, Gueye Ass Dia, definendolo «negro». Ripeto: sono notizie in attesa di verifica ed è quindi d'obbligo la massima cautela.

- sento il dovere di portare all'attenzione di quest'Assemblea quanto apparentemente accaduto nel corso di quella competizione. L'AIA ha avviato un'indagine e per bocca del suo presidente, Marcello Nicchi, e ha fatto sapere che chi ha sbagliato pagherà. Signor Presidente, i valori che lo sport porta avanti sono alti e condivisibili; in ragione e conseguenza di ciò, chi scende in campo ha enormi responsabilità. Mi riferisco all'esempio che calciatori, arbitri e addetti ai lavori sono chiamati a fornire ai nostri giovani e ai tanti appassionati. Mi auguro di no, ma se le notizie riportate trovassero conferma si tratterebbe di un episodio gravissimo da perseguire in maniera esemplare. Ripeto: attendiamo l'esito delle indagini. Sono episodi che rischiano di macchiare indelebilmente lo spirito e l'obiettivo delle competizioni sportive. Attenzione, cari colleghi: stesso discorso va fatto nell'altro senso. Tra i valori di cui parlavo e che lo sport ha il compito di tutelare e diffondere occupano un posto fondamentale lealtà e correttezza. Sarebbe quindi da condannare con egual fermezza un'eventuale montatura mediatica ad opera della società sportiva in questione o dei suoi rappresentanti. In quel caso, l'auspicio è che si provveda immediatamente a riabilitare la figura del direttore di gara coinvolto e che si prendano adeguati e pesanti provvedimenti nei confronti di chi ha gettato ombre su un'intera categoria e sul lavoro, spesso non facile, della classe arbitrale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

di un accentramento di impianti per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti: prima con l'inceneritore e poi con i maxi-impianti di discarica, di biostabilizzazione e di lavorazione e smaltimento di amianto. È notizia di questi giorni che nelle discariche Le Mate e Guarini di Cavallino sono stati rilevati e documentati da ARPA numerosi inquinanti pericolosi e cancerogeni, quali nichel, zinco, manganese e vari tipi di idrocarburi. Per i superamenti delle soglie segnalati negli ultimi dieci anni non risulta attivata alcuna procedura di caratterizzazione del sito, né si conosce quali siano i pozzi a monte e quali a valle della discarica, in base all'andamento della falda. Tanto per fare qualche esempio concreto, la discarica ex Saspi è una vera e propria bomba ecologica, misura 140.000 tonnellate di rifiuti velenosi tombati e non è mai stata bonificata, nonostante le richieste presentate alla Regione Puglia. Eppure, nella relazione tecnica redatta dagli incaricati della procura di Lecce, risultano riscontrate

e del completamento della piattaforma di biostabilizzazione RSU di Cavallino, sempre in località Guarini e Le Mate. E qui siamo all'assurdo, se consideriamo che con sentenza dell'aprile 2016, confermata dal Consiglio di Stato nell'ottobre 2018, il TAR di Lecce aveva ritenuto illegittimo il progetto dell'impianto, proprio perché in contrasto con le disposizioni che prescrivono una distanza minima dagli abitati e dai siti sensibili. Tale situazione complessiva è fortemente compromissoria per l'ambiente. Chiediamo, quindi, ai sindaci dei territori interessati di attivarsi in tal senso, anziché protestare al fianco dell'ennesimo tentativo di elusione; contestualmente, chiediamo alla Regione Puglia di mettere in atto finalmente delle misure preventive per salvaguardare la tutela della salute dei cittadini. Al territorio chiediamo di resistere, perché i cittadini non devono pagare le incurie e gli affari illeciti che si verificano